Le vittime, cinque donne e quattro uomini sono Nadia Benedetti, Claudio Cappelli, Vincenzo D'Allestro, Claudia Maria D'Antona, Simona Monti, Adele Puglisi, Maria Riboli, Cristian Rossi e Marco Tondat. Come sottolineato all'indomani della strage dal Presidente della Repubblica, erano nostri concittadini che operavano pacificamente, contribuendo alla crescita della società bengalese, sia attraverso attività imprenditoriali che mediante l'impegno nel volontariato e nel terzo settore. Insieme a loro, hanno perso tragicamente la vita altre undici persone di nazionalità giapponese, indiana, americana e bengalese. L'attacco terroristico di Dacca rappresenta l'ultimo di una lunga scia di attacchi sanguinari, che hanno visto anche il nostro Paese pagare un doloroso tributo di vittime innocenti. I carnefici sono spietati esponenti di un estremismo violento che, in nome del fanatismo religioso, cerca di minare i diritti dell'uomo e i valori della pacifica convivenza e della cooperazione tra i popoli e le culture. Analogamente all'attentato al Museo del Bardo di Tunisi, dove trovarono la morte quattro nostri concittadini, anche il massacro di Dacca si colloca nel quadro di una strategia terroristica volta a danneggiare quei Paesi di tradizione islamica che, attraverso il partenariato economico e culturale, instaurano relazioni con il mondo occidentale. In tale contesto, desta profondo turbamento la notizia secondo la quale gli attentatori sarebbero giovani bengalesi di buon livello culturale e di agiate condizioni economiche. Sarebbe la dimostrazione di come il fanatismo estremista riesca ad attecchire anche in fasce sociali non emarginate. Spetta a tutti noi, cominciando dalle istituzioni nazionali ed europee, reagire con fermezza a tale barbarie, sia attraverso gli strumenti della prevenzione e del contrasto al crimine terroristico, sia mediante la riaffermazione e la ferma difesa della libertà, della dignità umana, dell'eguaglianza, che costituiscono gli elementi fondanti della nostra civiltà. Il Senato della Repubblica si unisce, quindi, in un forte e sentito abbraccio al dolore delle famiglie e dell'intero Paese. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio.

il primo pensiero va alle vittime; a chi ha atteso loro notizie in quelle lunghe ore; a chi era così vicino da poter quasi vedere il proprio caro o la propria cara morire; a tutti quelli che volevano loro bene: questa è una morte che non si può spiegare, è una morte che non si può perdonare. All'indomani dell'attentato alle torri gemelle, gli Stati Uniti hanno dato il via alla più grande caccia internazionale al terrorismo, non senza errori, non senza tanti errori. i rappresentanti del terrorismo islamico, i taliban, al-Nusra, al-Qaeda, al-Shabaab, Daesh e tante altre sigle che abbiamo imparato a conoscere in questi anni siano solo e soltanto facce simili di uno stesso fenomeno criminale è profondamente sbagliato, che si tratti pur sempre di una minaccia circoscritta geograficamente, anche se in continua espansione, quasi un fronte del terrore sempre più vicino alle nostre porte o che il reclutamento o che il reclutamento e l'affiliazione ai gruppi jihadisti di nuove forze in Occidente avvenga nelle aree di disagio sociale proprio a causa dell'indigenza e della mancanza di prospettive, ad esempio nelle grandi periferie europee. Sono analisi che si dimostrano ogni volta parziali, superficiali e non esaustive. La notizia diffusa dal Ministro degli interni del Bangladesh, secondo cui gli autori della strage al ristorante di Dacca sarebbero membri del gruppo jihadista bengalese Jumatul Mujahedeen Bangladesh, tutti giovani di estrazione sociale - come ha ricordato lei, signor Presidente, un attimo fa - benestante, altamente istruiti, fra i quali essere miliziani jihadisti sarebbe una sorta di moda, ne è solo l'ultima conferma. Emerge chiara ed evidente una realtà diversa ma non nuova, nemmeno nella storia del terrorismo che ha colpito l'Italia nei cosiddetti anni di piombo: in questo caso, i miliziani non sono figli del disagio sociale né della povertà. Ci vantiamo di essere un popolo di grande e raffinata cultura, facciamo spesso appello a principi di solidarietà e di pace, di comprensione delle differenze; di essere in grado, meglio anche dei nostri alleati, di comprendere culture e realtà locali particolari, società organizzate su base tribale; abbiamo ritenuto di poter individuare le cause della diffusione del fanatismo religioso in Europa nella crisi culturale occidentale contrapposta al rinnovato fervore orientale, in grado di dare vecchie risposte a nuove domande, a nuovi bisogni. Ma non abbiamo capito che questa lettura da sola non spiega la proliferazione dell'estremismo anche nei Paesi islamici tradizionalmente laici. Un processo, dunque, socioculturale che va compreso a fondo, per spiegare anche come la mastodontica macchina della comunicazione messa in azione dal sedicente califfato sia così efficiente nel far circolare messaggi apparentemente tanto lontani dalle aspettative dei *millennial* italiani ed europei. Dobbiamo infine considerare che quest'analisi va ad innestarsi sulle dinamiche geopolitiche in atto nell'area mediorientale, che vedono tre conflitti sovrapporsi: la tradizionale contraddizione fra sciiti e sunniti; gli equilibri e gli interessi fra le grandi potenze regionali; la propagandata lotta contro gli infedeli occidentali. Serve dunque una risposta, una reazione alla minaccia terroristica, ferma, decisa, immediata; un'azione concreta, con ogni mezzo a disposizione, politico, diplomatico, militare e di *intelligence*, superando logiche di piccole contrapposizioni interne. Ma l'azione non può prescindere da una corretta analisi, prima di scoprire che anche i nostri figli sono alla ricerca di utopie e di ideali che non appartengono alle nostre radici culturali. Occidente ed Oriente nulla possono contro il nichilismo che, come unico collante, sembra coinvolgere e travolgere l'abbandono della consapevolezza della forza della propria storia. Teniamo a mente l'immagine di questi giorni che vede militari sciiti e sunniti pregare assieme nelle moschee della rioccupata (o liberata, a seconda dei punti di vista) Falluja, prima di tutto dobbiamo comprendere che i nostri primi alleati sono proprio coloro che all'interno del mondo islamico combattono contro il fanatismo e l'estremismo religioso. A questo riguardo, signor Presidente, vorrei chiederle - non so se altri Gruppi parteciperanno a questa richiesta - la

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso. Ebbene sì, lo dico da subito: mi scuso se non parteciperò a quelle commemorazioni di rito, basate sul *politically correct*, votate all'esaltazione del martirio, improntate su malposte basi di amor patrio, imbevute di un pietismo ipocrita, che si concludono sempre con ovvie banalità del tipo: l'odio non trionferà. Non indosso l'abito talare e lascio dunque le prediche a chi ne è avvezzo. Come parlamentare, invece, ho l'obbligo di seguire una religione prima di ogni altra cosa ed è la religione della ragione. Più ci penso e più mi convinco che non abbiamo modo migliore, non tanto per commemorare ma - vivaddio! - per onorare la memoria di questi connazionali trucidati dalla barbarie dell'Islam. Dobbiamo cioè domandarci, in modo laico, quale atteggiamento il mondo occidentale e in questo caso noi vogliamo avere nei confronti del mondo musulmano. «Se non ora quando?». Faccio mio questo motto tanto caro alla sinistra nostrana. Ebbene sì, questa è la domanda che, in modo imperativo, dobbiamo porci se vogliamo onorare le vittime e la nostra funzione. I nostri connazionali sono stati trucidati perché non conoscevano i versetti del Corano. Dopo i fatti di Parigi ho voluto leggerlo, giusto per capire se si trattava di differenze di religione o di differenze sociali e le conclusioni che ne ho tratto sono agghiaccianti, se penso all'atteggiamento di eccessiva comprensione e indulgenza che i "sinceri democratici" provano nei loro confronti. Valori fondanti della nostra civiltà, come la libertà e la democrazia, sono bestemmie per il Corano. Le donne sono incompatibili con il Corano i diritti umani sono incompatibili con il Corano. Insomma, il concetto stesso di civiltà, così come l'Occidente lo ha costruito, è incompatibile con il Corano e l'Islam è il Corano e il Corano è l'Islam. Allora, se così è - e a me pare che la terribile cronaca quotidiana si incarichi di confermarlo ogni giorno vieppiù - non è forse arrivato il momento Non è forse arrivato il momento di interrogarsi a proposito del controllo dei nostri territori? Non è forse arrivato il momento di ridisegnare la politica sull'immigrazione e i rapporti economici, compresi i Trattati, con tutti i Paesi musulmani? Vogliamo, cioè, privilegiare i valori di libertà e democrazia ancor prima dei valori economici? Mi chiedo e vi chiedo, ma iniziare con un'estensione del principio di reciprocità, internazionalmente riconosciuto, secondo il quale intanto ti faccio costruire una moschea, in quanto si possa costruire una chiesa nel tuo Paese, intanto sei libero di professare la tua religione nel mio Paese, in quanto sono libero di professare la mia nel tuo, può servire? O dobbiamo essere sempre disponibili a far calpestare ogni segno distintivo della nostra civiltà? Non c'è nessuno al mondo che difende la propria identità come i musulmani. Allora, nell'indignazione di pochi istanti può accadere che il padre massacri di botte la figlia perché ha osato indossare un jeans o che massacri di botte la moglie perché oggi gli va così, o che trovi offensivo il crocifisso nelle aule delle nostre scuole, o che si festeggi il Natale o la Pasqua o che sia da "cani infedeli" bere del Moscato o mangiare una costina di maiale. Ecco, noi siamo così per il Corano: siamo cani infedeli, ma sociologhi e intellettuali ci dicono che dobbiamo lavorare per l'integrazione. Ma leggessero il Corano, vivaddio! Maometto proibisce l'integrazione. E a proposito di sociologhi e intellettuali, come la mettiamo con questa strage di Dacca? I barbari assassini di questa carneficina non sono i miserabili delle *banlieue* parigine, gente che per ritorsione sulla mancata integrazione, condannata alla povertà, impugna il mitra e fa strage di cani infedeli. di Dacca sono i figli delle *élite* sociali del loro Paese, si sono formati nelle migliori scuole e università e hanno goduto degli agi che il loro ceto sociale aveva potuto loro garantire. Perdonatemi allora se uso con un po' di scherno le parole di Oriana Fallaci e mi chiedo dove sono oggi la sinistra al caviale, la destra al *foie gras* e il centro al prosciutto. Cosa ci diranno oggi questi esegeti del buonismo un tanto al chilo? Credo ci siano innumerevoli ragioni che ci obbligano a reagire. Abbiamo di fronte a casa una polveriera che si chiama Libia, alla quale la comunità internazionale guarda con algido distacco, snervante tatticismo e deprecabile lentezza. Bisogna iniziare ad occuparsene con grande intransigenza e determinazione. Abbiamo, o meglio sarebbe dire che subiamo un'ormai insopportabile immigrazione di stranieri, alla quale vanno date risposte diverse dalle semplicistiche ragioni attuali. Insomma, vanno maggiormente tutelati e affermati quelli che sono gli irrinunciabili interessi nazionali. E, per favore, risparmiatemi i giudizi puerili e sterili, volti ad affibbiare patenti di razzismo e xenofobia: sono sentimenti lontani anni luce dalla mia cultura. Prendiamo invece spunto dal grande esempio che ci viene dal fratello di una delle vittime, prendiamo esempio da padre Monti che, esaltando la sua missione evangelica, concede il perdono ai carnefici della sorella Simona. Esaltiamo allora anche noi la nostra missione, che è quella di garantire sicurezza e libertà ai nostri connazionali. Solo se faremo così avremo onorato la memoria degli italiani trucidati a Dacca.

Quella di Dacca è la giù grave strage jihadista di civili italiani dall'11 settembre 2001, quando 10 nostri connazionali morirono negli attentati alle Torri gemelle di New York. Un numero più alto di vittime italiane si è contato solo il 12 novembre 2003, quando nell'attentato di Nassiriya persero la vita 17 militari impegnati nel contingente italiano in Iraq. Si tratta del quarto episodio che coinvolge italiani nel solo 2016, dopo i fatti di Bruxelles, Tripoli e Burkina Faso, mentre nel marzo 2015 ricordiamo la strage al Museo del Bardo a Tunisi, che costò la vita a 22 persone, e a novembre la morte della studentessa ventinovenne Valeria Solesin nel massacro del Bataclan di Parigi. Le vittime si conoscevano tra loro: imprenditori del settore tessile, andavano spesso in quel ristorante che serve cucina mediterranea, forse per riassaporare i gusti del loro Paese, ma lì hanno trovato la morte, barbaramente torturati e uccisi a colpi di *machete*. È difficile per noi concepire una violenza simile: appare disumana, anzi lo è sicuramente. Come si fa ad accanirsi contro una giovane donna incinta e altre persone inermi? Questo è veramente inconcepibile. Da queste menti perverse ci separa una distanza siderale. Eppure, un manipolo di uomini sta tenendo in scacco il mondo con attentati continui, ma soprattutto facendoci vivere sotto una cappa di paura, colpendoci psicologicamente oltre che materialmente. La Lega Nord, il mio Gruppo, ormai da tanti anni porta avanti una battaglia, rimasta per molto tempo solitaria, a sostegno dell'identità dei popoli come unico strumento di difesa e di sostegno della nostra civiltà di fronte alle sfide mondiali e agli attacchi dichiarati da parte di altre culture. Soprattutto per questo motivo, forte è stato l'impegno del movimento nel denunciare la minaccia fondamentalista di matrice islamica, che è stata favorita e resa possibile dal diffuso atteggiamento multiculturale e buonista. La sfida fondamentalista non sarebbe infatti così impellente e pericolosa se non affondasse il colpo in un Occidente smarrito, che ha abbassato la guardia demograficamente, psicologicamente e spiritualmente, incapace di reagire perché assuefatto ad ideali di multiculturalismo e mondialismo necessari a una concezione economicamente fruibile della realtà, ma al prezzo di un relativismo senza uscita quanto riguarda valori, identità e tradizioni. Un relativismo che sabato sera ci faceva passare con una semplice pressione di un tasto del telecomando, dalle notizie di un massacro ad una partita di calcio. Eppure il mondo scoprì l'esistenza del Bangladesh nell'agosto del 1971, quando alcuni grandi artisti, tra cui Bob Dylan ed Eric Clapton, salirono sul palco per un concerto di beneficenza. Fu una delle prime idee di globalizzazione: c'era la musica, c'erano i buoni sentimenti, c'era una raccolta di fondi per i bambini che morivano di fame in quella minuscola scheggia di continente indiano, stremata dalla carestia e dalle guerre civili, che avevano fatto, tra le altre cose, tre milioni di morti e decine di milioni di profughi. Le vittime italiane della strage di Dacca erano tutte troppo giovani per avere memoria di quel concerto. Il loro Bangladesh era un'altra cosa, una seconda patria, dove fare impresa fidando sul buon tasso di crescita, sulla docilità dei lavoratori del settore tessile e su una illimitata manodopera e questo in nome della possibilità di vivere in un villaggio globale, in cui anche l'attrezzata società diventa risorsa e attrae investimenti. Attenzione alle piccole fabbriche e al lavoro: questi erano i nostri concittadini. Ma il Bangladesh, signor Presidente, non è l'unico Paese al di fuori dei confini europei e non in guerra dove gli italiani potrebbero essere nel mirino del terrorismo. Sono circa 35.000 le imprese sparse sparse in tutto il Nord Africa e nei Paesi arabi. Se quello è stato un attacco agli italiani, dovremo avere la massima attenzione, signor Presidente, perché a volte si hanno estremi danni anche senza avere attentati in casa. Vede, signor Presidente, ai kamikaze che muoiono combattendo contro i nemici dell'Islam poco importa se producono solo stragi di innocenti: con le loro azioni suicide acquistano il diritto di entrare in Paradiso con la qualifica di martiri. Mi spiace, signori, voi per me non siete martiri: siete solo brutali assassini, e pure vigliacchi. Voi in Paradiso non metterete piede. Adele, Marco, Claudia, Nadia, Vincenzo, Maria, Cristian, Claudio e Simona: per voi le porte del Paradiso sono spalancate. *(Applausi

la strage di Dacca ci ha messo di fronte ad un dolore dinanzi al quale ci siamo trovati impreparati ed assuefatti nello stesso tempo. Cosa intendo dire? Intendo dire assuefatti e impreparati, perché nel giorno della tragedia i nostri *media*, le nostre televisioni e le radio non sapevano come gestire, ad esempio, la presenza della partita di calcio della nazionale, a fronte di un lutto così immenso. Nel giro di cento ore sono avvenuti attentati tragici e mostruosi (è difficile trovare gli aggettivi adatti): Istanbul, Dacca, Baghdad. Eppure, nello stesso tempo, corriamo il rischio che questo non determini un incremento della nostra consapevolezza di fronte al male che mostra il suo volto più orrendo e che perdiamo il significato del dolore bruciante che, nella lontana Dacca, ci siano nove italiani uccisi con indicibili crudeltà perché non conoscevano a memoria il Corano. Un rito blasfemo, osceno, degno di una guerra senza quartiere. Di fronte a questa distruzione della ragione, come dovrebbe rispondere il mondo della democrazia e della civiltà occidentale? Quello che ci si aspetta è certo la compattezza di un fronte della razionalità e del buon senso contro la barbarie. Una compattezza di principi. Una compattezza, se necessaria, di collaborazione militare, di *intelligence*, di prevenzione e di solidarietà. Insomma la difesa della propria identità, che ha di fatto guidato il mondo democratico nel suo difficile cammino verso pace e sviluppo. Eppure tutto questo non sarà possibile se non impareremo a chiamare le cose con il loro nome. Non capire che la battaglia contro il terrorismo dell'ideologia islamista è un compito comune può solo favorire le forze della irrazionalità, il rancoroso nichilismo degli jihadisti benestanti del Bangladesh, il non senso della vita, il rancore nei confronti della materialista società mondializzata, che spingono verso un approdo dove nichilismo e giustizialismo si fondono: è in nome di una presunta giustizia divina che i terroristi si sono sentiti legittimati a uccidere e a far soffrire le loro vittime. Teste e cuori vuoti, a Dacca come a Molembeek, sono più pericolosi di stomaci vuoti. E il prendere in ostaggio il nome di Dio per il proprio progetto di potere sarebbe forse valso anche stavolta agli assassini l'impunità,

dal sacrificio del giovane Faraaz Hossein, che, a testimonianza di cosa voglia dire comprendere la grandezza di Dio, ha sacrificato la propria vita per obbedire alla voce della sua coscienza e stringersi alle amiche musulmane vestite in modo troppo occidentale e agli infedeli italiani e giapponesi con cui condivideva un di più di umanità vera che non sarà mai dei suoi carnefici. Stringiamoci allora anche noi, alle famiglie delle vittime, «stringiamoci a coorte», come recita il nostro inno nazionale, perché nel nostro Paese la coscienza prevalga sull'indifferenza. E stringiamoci anche - non ho tema di dirlo su questa materia - al fianco del nostro Governo, perché con paziente determinazione contribuisca, nella comunità internazionale e di fronte agli scenari di guerra che perdurano, al prevalere della razionalità della politica e dei nostri ideali, in nome di una Italia che sappia essere unita nel combattimento che la storia gli affida. mi auguro che ascoltando questo suggerimento si presenti al più presto in Aula il Ministro degli affari esteri, che voglia condividere con noi non solo le preoccupazioni, ma anche le strategie perché questa guerra si vinca. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto a nome del Gruppo di AL-A esprimo sentimenti di cordoglio per le vittime

colpendo civili innocenti, imprenditori e lavoratori che a migliaia di chilometri dal proprio Paese cercavano una risposta alla globalizzazione dei mercati. Bene hanno fatto le massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, a rivolgere un appello a tutto il popolo italiano a ritrovare quell'unità indispensabile in questi momenti, che deve servire fortemente a creare le condizioni per reagire nella giusta maniera di fronte a fatti così efferati. Ma non è solo è Istanbul, è Bagdad; è una guerra infinita diversa dalle solite guerre, ma proprio per questo più insidiosa e difficile da combattere. Ora non è il momento dei distinguo, dei facili *j'accuse* contro coloro che per appartenenza geografica vivono anche sul nostro territorio. Non è il momento di chiudersi in nazionalismi esasperati che servono invece a creare le condizioni perché venga meno quell'unità per contrastare il terrorismo e combatterlo, affrontare le sfide che riguardano il nostro Occidente. È il momento in cui, come dimostrano i fatti di Dacca, il terrorismo non trova più quelle giustificazioni sociologiche della retorica post-marxista

Oggi non è il momento di un coro sulla mancata sicurezza, sui controlli che saranno stati pochi o omessi e sulla sottovalutazione del pericolo. «Si sarebbe potuto fare di più»: è così che si dice spesso; ma oggi non è il momento

Martiri sono i nove italiani uccisi in quel modo e non le persone che li hanno ammazzati. Coloro che li hanno uccisi sono terroristi islamici, non vi è dubbio, perché ammazzano citando e nel nome di Allah. Attenzione però, perché non direi che sia l'Islam che trae profitto da questi assassini, piuttosto direi che l'Islam ne è l'ostaggio, è il terreno di questa conquista.

superare la censura interna e il disinteresse generale che c'è nei confronti del Bangladesh, colpendo con uno schiaffo al volto la classe dirigente islamica del loro Paese, cioè i loro stessi padri, come è stato detto e notato. Contemporaneamente, un altro attentato ammazzava a Bagdad 25 bambini sciiti e oltre 200 persone. Islamici che ammazzano musulmani. Poco prima c'era stato l'attentato a Istanbul: un messaggio da parte di *killer* che venivano dall'ex Unione sovietica all'ex amico del Daesh,

presuppongono due cose, entrambe profondamente sbagliate. La prima è che sia possibile alzare un muro che ci protegga da un virus che si presume venga dall'esterno.

tutto sommato per noi non va male. Questa è la politica dell'imperialismo in Medio Oriente e nelle terre dell'Islam. Non è così: se gli islamici si scannano tra di loro, ci prendono in ostaggio e lo fanno a Dacca, a Istanbul e anche al Bataclan di Parigi. Dobbiamo sapere ciò e anche che difendere e sostenere i cosiddetti Stati arabi moderati (che spesso sono corrotti e responsabili di aver pagato quegli *imam* integralisti che hanno diffuso anche in Occidente la teoria della *jihad* a vita)

Guardate che lo *jihad* wahabita è una risposta semplificata e molto efficace alla mondializzazione. Non a caso se ne cominciò a parlare al tempo della prima mondializzazione, con l'illuminismo, l'imperialismo inglese e le guerre napoleoniche. Questo *jihad* wahabita semplifica oltre modo il Corano e l'Islam e nega ogni possibile mediazione; nega la grande storia dell'Islam: Avicenna, Averroé, l'Alhambra e potrei continuare. continuare. Nega persino il monumento al profeta perché anche questo indebolisce l'aspetto di totale sottomissione al dio, che poi significa sottomissione al califfo, cioè al capo temporale e guerriero, che è l'elemento fondamentale di questo virus che si insinua

a Orlando ve lo ricordate? Probabilmente si trattava di un giovane americano, anche con pulsioni omosessuali, che ha sterminato una comunità di omosessuali. Quanto successo a Saint-Denis l'avete dimenticato? Avete visto le foto di quel signore con la moto e le ragazze nude che poi ha fatto la strage al Bataclan? Il virus è dentro di noi e far finta che non lo sia, pensare di poterlo isolare senza combattere la mondializzazione dal volto non umano con una mondializzazione dal volto umano sarebbe un errore gravissimo e imperdonabile.

raccontare cos'è il Bangladesh, che c'è una guerra della nostra alleata e amica Arabia Saudita nello Yemen e che questa guerra è come una ferita purulenta che provoca altre Oggi difendere i diritti in tutti i Paesi e quindi non avere degli atteggiamenti corrivi nei confronti di una parte dell'Islam cosiddetto moderato è fondamentale per isolare e battere questo fanatismo nel nome

altri discorsi mi sono sembrati più deboli e meno centrati sulla vera ragione della sfida. Concludo dicendo che, se dobbiamo veramente onorare i martiri italiani a Dacca, la cosa da fare è avere capacità di analisi schiette, franche e anche di essere conseguenti. A questo punto, chiedo con forza, a nome di tutto il Gruppo, il dibattito in Assemblea con il Presidente del Consiglio.

Noi dobbiamo esprimere in questo momento - che non è quello dell'analisi approfondita - la solidarietà alle famiglie e unirci simbolicamente con il sentimento forte di quest'Aula

(come abbiamo visto nei giorni scorsi nel Kurdistan iracheno ad aiutare le donne yazide o i cristiani scappati); ai militari che rappresentano il meglio della nostra italianità e che sono lì impegnati come strumento fondamentale della politica estera. ISIS, Al Qaeda, gruppi terroristici di tutti i tipi e le risme sono all'attacco è giusto che da questa vicenda del Bangladesh traiamo anche delle conclusioni per evitare grandi errori di sottovalutazione o di sopravalutazione. che nei giornali italiani si esprime grande interesse sul fatto che questi criminali fossero e sono figli dell'alta borghesia di quel Paese. Ma Bin Laden chi era, se non il prodotto della sottospecie della casa reale saudita che nella sua lotta per cambiare gli equilibri nel grande regno saudita traeva spunto e utilizzava anche persone di ceti infimi come manovalanza del terrore spietato che aveva messo in essere? Dunque, io credo che si ripropone la drammatica domanda che ci facciamo tante volte all'indomani delle stragi. La risposta non è quella di identificare in una classe sociale la figlia di queste vicende; purtroppo le classi sociali sono le più disparate, e il terrorismo è un grande male unificante. Vorrei dire anche che un'altra domanda che si ripropone sempre è quella se ci sia una guerra di religione in atto. Consentitemi di concludere solo volendo ancora una volta dire: fermiamoci. I musulmani nel mondo sono miliardi, i cristiani nel mondo sono miliardi; evitiamo noi stessi di cadere nella trappola di chi, con quella richiesta di evocazione del Corano, dimostra in modo chiaro e lampante il proprio disegno: creare nel mondo una guerra impostata su basi religiose. È esattamente quello che noi, in nome della nostra civiltà e della nostra concezione della libertà religiosa dobbiamo rifiutare. Nessuna guerra si può fare in nome di Dio: così ci disse Giovanni Paolo II proprio in Parlamento. Bene, noi da quell'evocazione di un grande Papa traiamo un senso civile comune che unisce tutta quest'Aula. Non c'è una guerra di religione in atto, c'è il tentativo di leggere in modo distorto alcune pagine del Corano da parte di chi utilizza l'Islam o vuole utilizzarlo per dividere l'umanità. Ma in realtà obiettivi non solo cristiani. Questa volta sono caduti gli italiani, ma a Tunisi, in Iraq, in Arabia Saudita, cadono islamici, perché questo terrore non ha confini di appartenenza, di nazionalità, di religione e colpisce tutti in modo indiscriminato. Il vero problema,

tra chi di questa civiltà si vuole fare portatore dei suoi valori ed anche delle sue contraddizioni (perché no, siamo in una civiltà piena di contraddizioni), e chi la vuole abbattere. Penso che non che non siano caduti invano i nostri connazionali: è una tappa di una battaglia che sarà lunga, di una lotta che si deve fare senza quartiere, avendo la consapevolezza che l'Italia è in prima linea. Qui non c'è nessuno che può dichiararsi fuori da questa guerra, perché questa guerra al di là delle nostre volontà ci coinvolge. L'Italia è in prima linea come gli altri Paesi, e mi piace concludere evocando Faraaz Hossain, il giovane che si è sacrificato per non lasciare sole le sue compagne che avevano la sua stessa religione, e per non lasciare soli i nostri connazionali. È l'esempio straordinario di un ragazzo meraviglioso che aveva concezioni religiose diverse dalle nostre, ma che con noi è unito dal senso di un'appartenenza a un destino comune.

probabilmente ogni relatore ha una parte di ragione, perché forse i motivi sono tanti e non c'è un unico motivo che possa spiegare questi atti così efferati, che possa spiegare le origini e il dispiegarsi del terrorismo.

cioè la realtà degli organismi esterni penetrati in determinate regioni per accaparrarsi le materie prime; in buona sostanza, sto parlando di organismi multinazionali. Ricordiamo che anche Papa Francesco nella sua ultima enciclica ha detto chiaramente che le multinazionali arrivano spesso devastando un territorio e lasciando dietro di loro una scia di devastazione.

Mi domando, altresì, se una di queste cause non sia la deregolamentazione del mercato finanziario accaduta negli ultimi decenni; una deregolamentazione che ha letteralmente sguinzagliato il potere finanziario, amplificato anche dall'avvento dell'informatica, che ha esasperato le velocità di transazione, le possibilità di moltiplicazione del denaro elettronico in circolazione e l'introduzione di una serie di nuovi strumenti dovuti alla mancanza di regole. Ciò ha esagerato la forza della cosiddetta leva finanziaria e, quindi, moltiplicato il denaro e il fatto che questo potere finanziario, in molti casi, sfrutta

oppure gli investimenti sull'economia e sulla finanza virtuale, che amplificano ulteriormente la situazione di mancanza di democrazia. Certamente, uno dei motivi può essere anche quello della religione, ma storicamente sappiamo che la religione è spesso un paravento per difendere gli interessi economici. Qui probabilmente siamo in presenza dell'ennesimo atto di *divide et impera*: io creo confusione nella regione, amplifico le differenze e i motivi di odio reciproco in maniera da poter sfruttare più comodamente le risorse sia di materie sia di materie prime e di manodopera che quella regione mi mette a disposizione. Vorrei concludere con un appello. Come politici, sappiamo perfettamente che dovremmo agire a livello legislativo per per ridurre ed eliminare tutte queste cause. Io faccio però un appello anche ai cittadini che ci ascoltano, che non sanno che il denaro che depositano negli istituti di credito viene utilizzato, con una leva finanziaria di 500 a 1, nella finanza virtuale e speculativa,

che non rovina le persone che lavorano in quella economia. Quindi, noi come legislatori abbiamo il dovere di minimizzare ogni causa possibile, ma mi appello anche ai cittadini perché anche loro possono fare moltissimo; il mare è formato da tante piccole gocce e, a causa della leva finanziaria, anche il potere del singolo cittadino è molto più elevato di quello che egli ritiene di possedere. Quindi, mi appello anche ai cittadini affinché diano

debbo dire che fatico a trovare parole adatte ad esprimere il grande dolore delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico per la morte di nove italiani assassinati lontano dalla loro Patria. Abbiamo letto tutti le loro storie: erano nove italiani innocenti, perbene, persone pacifiche, grandi lavoratori; italiani che hanno fatto onore all'Italia nel mondo, che hanno fatto conoscere il nostro Paese, lo hanno fatto rispettare e lo hanno fatto anche amare. Il loro assassinio è molto più di un atto di violenza, di efferata crudeltà, di sanguinario e atroce cinismo: è un atto vile, codardo. Questi continui assassinii di donne, uomini e persino bambini, tutti innocenti, uccisi per fare spettacolo della morte, per avere i titoli dei giornali, per richiamare l'attenzione delle opinioni pubbliche, fanno tutti ribrezzo e sono quanto di peggio possa dare la natura umana quando si ammala così gravemente. La morte ingiusta di nove italiani buoni si iscrive in una drammatica e lunghissima sequenza di omicidi, di stragi, di vere e proprie mattanze che ormai da anni, con violenza e frequenza sempre maggiori, per mano del cosiddetto terrorismo islamista, stanno insanguinando il mondo, tutto il mondo: dal continente americano all'Europa, dall'Asia al continente africano. C'è un evidente intento politico dietro a tanto orrore. C'è la volontà insensata di colpire sia l'Occidente sia la vastissima parte del mondo islamico che non accetta la violenza e il terrore. Sappiamo quanto sia difficile e lunga la lotta al terrorismo. Lo è stata negli anni Settanta e Ottanta in Italia, lo è ancora di più ora che ha assunto un'incontrollata dimensione globale, ma non possiamo accettare che questa barbarie continui; non possiamo accettarlo perché abbiamo il dovere di difendere donne e uomini innocenti. Non possiamo accettarlo anche perché nella storia dell'umanità una violenza terroristica così sanguinaria e così diffusa è sempre stata l'anticamera della guerra, di una guerra che oggi sarebbe spaventosa, che non si capisce neanche contro chi sarebbe, di una guerra che il mondo deve impedire con ogni mezzo e a qualunque costo. Lo ripeto, chi sta seminando il terrore nel mondo ha un'intenzione chiara e dichiarata: vuole sempre più distruzione, sempre più morti. Vuole che non ci si senta al sicuro da nessuna parte, che si tema di essere colpiti ovunque. L'Italia deve ringraziare le sue forze di polizia, le sue Forze armate, la sua *intelligence*, la sua magistratura e la sua diplomazia. Sono gli uomini e le donne che, con grandissima professionalità e sacrificio, stanno proteggendoci da un pericolo reale che opera nascosto, mimetizzato, codardo e che colpisce sempre a tradimento. Dobbiamo aiutare le forze di polizia, le Forze armate, l'*intelligence*, la magistratura, la diplomazia; dar loro le risorse, le dotazioni e gli uomini di cui hanno bisogno perché la sicurezza nazionale è nelle loro mani.

ma noi senatori, noi parlamentari dobbiamo chiederci cosa ciascuno di noi può e deve fare per aiutare l'Italia e l'Europa a difendersi meglio. Io credo che il nostro primo dovere sia quello di mostrare un Paese unito; almeno unito sui grandi temi della sicurezza, un Parlamento dove si discute ma non si insulta, un Parlamento dove maggioranza e opposizione non si spacchino sulla difesa dei principi fondamentali della pace e sulla difesa della vita dei cittadini. Uno degli obiettivi dei terroristi è dividerci: uccidono anche per questo, per alimentare le divisioni nelle democrazie occidentali, per creare il *caos*, per farci saltare i nervi. Se vogliamo rispondere alla violenza con la forza della nostra democrazia (e la nostra democrazia deve in questo caso dimostrare la sua forza), mostriamo loro la nostra capacità di coesione e la nostra unità nazionale.

Ai familiari delle vittime del barbaro attentato in Bangladesh vorrei esprimere qui in Aula, a nome del Governo, il più sentito cordoglio e la stretta vicinanza al loro profondo dolore. È un dolore che ci accomuna tutti e che ci farà stringere tutti in un ideale abbraccio nel momento in cui questa sera, all'aeroporto di Ciampino, accoglieremo le salme dei nostri nove connazionali. Questa mattina il vice ministro Giro è atterrato a Dacca per accompagnarle nel viaggio di ritorno a Roma, dove saranno ad attenderli il presidente Mattarella e il ministro degli esteri Gentiloni.

Sono state barbaramente uccise persone la cui volontà - mi pare evidente - era di amicizia e non di ostilità, di intesa e non di divisione. Purtroppo quello di Dacca costituisce il più grave attentato ai danni dei nostri connazionali dopo quello avvenuto a Nassiriya. Non è che l'ultimo, in termini di tempo, di tanti tragici avvenimenti che hanno segnato la vita degli ultimi anni e che hanno provocato una lunga scia di vittime innocenti, italiane e non. Oggi è di nuovo il momento di piangere la perdita di vite umane, come quelle di Bruxelles, Istanbul, Ankara, Tunisi, Parigi, in Siria e in Iraq e nelle altre aree di crisi. Penso che non dobbiamo, però, cedere allo sconforto e alla paura, né alla rassegnazione; soprattutto non dobbiamo tradire il senso profondo dei nostri valori. La nostra reazione deve essere tanto forte quanto l'impatto emotivo che hanno avuto in noi le immagini del ristorante di Dacca, dell'aeroporto di Istanbul, del Bataclan di Parigi. L'odioso attentato in Bangladesh ci impone di non arretrare di un millimetro nella lotta contro il terrore e ci deve spingere a rafforzare ulteriormente tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare il terrorismo e i suoi efferati intenti. Ovviamente non parlo solo di sostegno a chi combatte Daesh sul campo, ma anche di rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello internazionale a tutti i livelli, cogliendo - credo - l'evoluzione del fenomeno, che certo non è più determinato solo da condizioni sociali, piuttosto da contesti ambientali e di area globali. La distorsione della religione a scopi di dominio: questo è l'intendimento e l'uso che se ne fa. Dobbiamo isolare il terrorismo fondamentalista dentro la realtà del mondo islamico e dobbiamo farlo chiedendo alle comunità islamiche nei nostri Paesi e ai Governi dei diversi Paesi islamici di impegnarsi con noi al massimo livello possibile. Lo dobbiamo alle vittime dell'attentato. Lo dobbiamo ai nostri figli, che vogliamo possano crescere in un mondo sicuro e non pervaso di odio e terrore. Lo dobbiamo ai nostri valori, alla tolleranza, al rispetto per l'altro, al rifiuto della violenza, a tutti quei principi per i quali abbiamo lottato nel corso dei secoli e ai quali non vogliamo rinunciare. È tempo davvero di una nuova e appropriata resistenza per sconfiggere gli usurpatori del nostro tempo: gli usurpatori di libertà, che colpiscono ogni civiltà, ogni comunità e ogni religione. Il Presidente del Consiglio ha lanciato in questi giorni un forte appello a tutte le forze politiche e sociali per vivere insieme questa pagina di dolore, di cui in questa sede è stata data ampia testimonianza, davanti alla tragedia dell'estremismo radicale. infatti, che crediamo «sia il momento in cui l'Italia dia un messaggio di dolore e compassione. Piangiamo lacrime di solidarietà e di cordoglio, ma è anche il momento di lanciare un messaggio di determinazione: l'Italia non arretra davanti alla follia di chi vuole disintegrare la vita quotidiana».

Signor Presidente, come ha ricordato, il disegno di legge che oggi è al nostro esame è già stato esaminato e approvato in prima lettura al Senato, devo dire parecchio tempo fa. Torna oggi in Aula per un terzo esame dopo che la Camera dei deputati ha approvato un testo che contiene una serie di modifiche, rispetto a quello originario approvato da noi, che configurano un impianto solo in parte diverso, ma che a mio avviso confermano la validità della prima scelta della nostra Assemblea e anche molte delle caratteristiche fondamentali che volemmo imprimere al provvedimento.

dunque soffermarmi brevemente su alcune caratteristiche che dicono come questo provvedimento, nel suo complesso, sia qualcosa di estremamente utile per il nostro mondo del comparto primario. Esso costituisce un contributo molto significativo: ne fa fede anche la grande attesa che i nostri agricoltori da tempo ci hanno segnalato perché il Parlamento vari definitivamente il provvedimento Il testo affronta profili che rivestono una rilevanza fondamentale per il comparto sia sotto l'aspetto istituzionale, che sotto quello economico. Voglio ricordare brevemente che i temi fondamentali su cui interveniamo sono quelli della semplificazione - mai come oggi necessaria in tutti i comparti produttivi, a partire da quello agricolo e riordino di molte normative, il tema dell' imprenditoria giovanile, il riordino degli enti e delle agenzie vigilati dal Ministero, lo sviluppo delle imprese, la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura e il sostegno alla filiera corta e all'agricoltura biologica.

in vari settori, tra cui l'adozione di un codice agricolo e di eventuali appositi testi unici, e l'adozione di norme sul ricambio generazionale in agricoltura, che ovviamente si prefiggono di favorire l'ingresso dei giovani nel comparto e l'avvio e la prosecuzione di nuove imprese. Esso contiene ancora disposizioni di sostegno all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, settori in grande espansione e di notevole interesse per i consumatori. Inoltre, vi sono anche specifiche disposizioni su singoli settori merceologici di particolare interesse per il nostro Paese: cito tra gli altri il pomodoro, il riso, il miele e i prodotti apistici, la birra artigianale, i funghi, i prodotti ittici, la già citata pesca e l'acquacoltura. A questo punto vorrei anche sottolineare - signor Presidente, mi sarà permesso - i lavori svolti nel corso dell'esame in Commissione. È stato anche questa volta un dibattito approfondito, che ha permesso di prendere in esame tutti i punti del provvedimento e ha consentito a molti di sottolineare il valore stesso del provvedimento come quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario, attraverso misure che consentiranno di dare un ulteriore impulso al settore agricolo. che si possa dire che dalla collaborazione tra Senato e Camera dei deputati, sia pure in un lasso di tempo che molti (tra i quali anche io) avrebbero desiderato fosse più breve, siamo giunti a un testo che, dopo gli ampi spazi di approfondimento garantiti dalle diverse letture, appare arricchito di nuovi fondamentali contenuti rispetto alla sua formulazione originaria. Vorrei sottolineare come l'esame in Commissione abbia consentito di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche molto importanti, le quali sono a loro volta suscettibili non solo di un utilizzo immediato, ma anche di costituire un ulteriore utile spunto di riflessione e di approfondimento anche in prospettiva per ulteriori futuri interventi normativi. Fa fede di questo lavoro di Commissione anche l'ampia presenza di ordini del giorno, nei quali la Commissione ha voluto sottolineare fatti nuovi sui quali stimolare l'azione del Governo e sottolineo che molti di questi ordini del giorno sono stati valutati positivamente dal Governo e accolti, come sarà chiaro quando passeremo in fase di votazione. Tra i temi trattati in questo nostro lavoro desidero ricordare i profili come la proprietà coltivatrice, la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, la zootecnia delle aree montane, la garanzia al credito per le aziende agricole, la registrazione telematica dei contratti di rete, oltre a numerosi interventi nel settore lattiero-caseario e ancora il regime giuridico relativo a determinati rifiuti agricoli, ai comparti frutticolo e agrumicolo. Insomma, ritengo veramente che si possa dire che il testo che giunge al nostro esame e al voto di oggi sia un legittimo frutto di una riflessione approfondita che ha permesso una definizione meditata dei contenuti e che ha visto il contributo e un'ampia convergenza delle forze politiche. Citavo numerosi ordini del giorno; mi sia permesso sottolinearne tre da me presentati. Il primo è relativo al regime di sfalci e potature, che ha presentato alcune criticità ad un esame più più approfondito rispetto a quello che la Camera dei deputati aveva potuto realizzare. L'ordine del giorno invita il Governo a monitorare gli effetti della norma e a valutarne un'eventuale modifica qualora sia foriera di incertezza applicativa o di disparità di trattamento. Sottolineo ancora altri due ordini del giorno che riguardano il comparto della birra e il settore agrumicolo. Mi avvio alla conclusione. Ho ricordato già prima come i nostri agricoltori attendano da tempo questo provvedimento. Auspico quindi che il Senato possa approvare definitivamente il provvedimento stesso, che rivelerà i suoi influssi positivi non soltanto sul comparto dell'agricoltura, ma anche - io penso - sull'intera economia nazionale, di cui il settore primario rappresenta un sostrato imprescindibile. Penso che possiamo definire questo collegato agricolo come un tassello ulteriore, che va ad aggiungersi alle leggi in materia di agricoltura già approvate definitivamente nel corso della presente legislatura. Sono parecchie, colleghi; abbiamo lavorato intensamente, tra Senato e Camera, su questi temi. Cito, tra le altre, la legge sull'agricoltura sociale, la legge sulla tutela della biodiversità agraria e alimentare, nonché la conversione del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, oltre ai profili di competenza di leggi più ampie. Voglio concludere realmente, signor Presidente e colleghi, sottolineando come sia proprio di queste settimane il dato che ci consegna i risultati in crescita dell'agricoltura italiana in questi trimestri, in particolare nel Sud. Questi dati positivi ci dicono di un risveglio del mondo dei nostri coltivatori e di un nuovo interesse delle giovani generazioni. E credo che ci permettano anche di dire, con soddisfazione, che forse la nostra azione legislativa non è stata inutile, ma ha dato qualche contributo. Quindi intendiamo consegnare questo ulteriore frutto del nostro lavoro a tutti gli operatori del settore primario, perché possa essere di aiuto al loro lavoro. e colleghi, il disegno di legge collegato agricoltura diffusamente delega al Governo ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare

un grande impegno propulsivo e la volontà di rilancio di una dinamica economica e sociale del Paese, attraverso una produzione di riforme quadro e di settore e la messa in campo di interventi finalizzati ad incentivare la propensione imprenditoriale, soprattutto dei giovani, e anche il coinvolgimento collettivo di ultrasessantacinquenni e pensionati. Un obiettivo che si propone di favorire la necessaria osmosi tra la politica e l'universo articolato del sociale. Per favorire lo sviluppo del Paese del Paese reale è necessaria una capacità inventiva e processi vincenti: giovani che tentino la strada delle *start-up* in agricoltura e nell'agroalimentare, imprese che investano in innovazione e in *green economy*, collaborazione e cooperazione intergenerazionale, capaci di favorire gli scambi di conoscenze e competenze, di saperi nuovi e antichi tra le varie fasce di età. I territori dell'impresa agricola diventano luoghi, laboratori, *hub* di relazionalità, di integrazione delle differenze nella nostra quotidianità. Il *made in Italy* ritrova questi fondamenti nell'integrazione tra gastronomia e filiera agroalimentare, nell'integrazione tra agricoltura, ambiente, turismo e cultura. Il provvedimento dunque è di ampia portata innovativa e viene approvato dopo un lungo esame, in cui è stato modificato, come è stato ben sottolineato dal relatore poc'anzi. Alcune sue parti, inserite in decreti d'urgenza, sono quindi legge dello Stato. La finalità del provvedimento, che si inserisce nella *road map* del Governo, è principalmente quella di liberare il mondo agricolo dall'ossessione normativa, di sburocratizzare, di rendere più rapido, efficiente ed efficace tutto il sistema dei controlli. Sulla semplificazione e i controlli, appunto, mi pare importante segnalare la riduzione dei tempi per la pubblica amministrazione (sessanta giorni) per rispondere alle richieste presentate dai centri di assistenza agricola; l'eliminazione del fascicolo aziendale per i piccoli produttori di olio (meno di 350 chili annui); nuove norme sui requisiti di etichettatura e confezionamento dei derivati dalla trasformazione del pomodoro; introduzione di sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica; il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal MIPAAF; la riorganizzazione di AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; il riordino del sistema dei controlli; la razionalizzazione delle società di Agecontrol SpA; l'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali, nonché la destinazione delle risorse risparmiate all'internazionalizzazione del *made in Italy*: tutto ciò potrebbe fare la differenza per il futuro del sistema dell'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi comunitari nella direzione di un miglioramento della qualità dei servizi alle aziende agricole, che - voglio sottolineare - stanno attraversando un periodo di lenta e faticosa ripresa trasversale un po' in tutti i comparti. Mi preme evidenziare la grande conquista di civiltà che comporta l'inserimento negli statuti dei consorzi di tutela del principio di equilibrio di genere negli incarichi. Lo statuto dei consorzi deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri, appunto, questo equilibrio. Dopo un lungo periodo di crisi, quindi, che ha visto la chiusura di imprese, l'abbandono di terre, la chiusura delle stalle, lo svilimento del ruolo delle imprese agricole, vengono dalle nuove misure già in atto, incluso il collegato, un nuovo impulso al nostro Paese, una spinta all'economia, un supporto alle piccole e medie imprese, un incentivo agli accordi di filiera, oltre che all'innovazione tecnologica e informatica, all'agricoltura di precisione e al trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario. Salto una parte del mio intervento, che consegnerò agli atti, per non rubare tempo agli altri colleghi, ma voglio sottolineare ancora qualcosa. È importante - a mio avviso - la previsione di criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni degli sgravi fiscali a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne pensionato e del giovane imprenditore agricolo.

tra agricoltore più anziano e agricoltore più giovane, con forme di compartecipazione agli utili di impresa e riconoscimento del diritto di prelazione per i giovani in caso di vendita di terreni oggetto oggetto del rapporto di affiancamento tra le due generazioni. Le forme agevolative a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli costituiscono un ulteriore significativo elemento di non poco conto. Una politica agricola nazionale, dunque, che contribuisca ad arricchire le pagine del *made in Italy* non può essere restia all'innovazione né avara di investimenti, ma deve

per l'ottimizzazione dei processi produttivi. Dai miei incontri con gii istituti agrari, ma pure dall'audizione in Senato in Commissione Agricoltura della presidente della rete degli istituti professionali e tecnici agrari, emerge questa riflessione, la necessità di mettere in grado i giovani di confrontarsi con strumenti e tecnologie innovative,

il lavoro, comporta quattrocento ore di operatività concreta in azienda. E questa è una condizione necessaria per tutti gli studenti in generale, ma essenziale a maggior ragione per il mondo agroalimentare. È, quindi, ancor più ragionevole e legittimo prevedere un potenziamento e un aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che devono essere all'avanguardia in quelle aziende che, soprattutto come quelle annesse alle scuole, sono parte strutturale e intrinseca dell'istituto stesso. Segnalo di aver presentato su questo tema un ordine del giorno per tentare di far dotare gli istituti

quando l'allora presidente del Consiglio dei ministri Letta presentò il provvedimento. Tra l'altro, leggendo l'elenco dei Ministri che lo sottoscrissero, alcuni nomi non si trovano più neanche nell'elenco del telefono.

Quindi, alla fine, le cosiddette riforme del Governo, nel momento in cui non producono risultato, non sono più sostenibili e diventano addirittura degli orpelli che appesantiscono ancora di più il lavoro di chi, in questo caso, si occupa di agricoltura. Il passare del tempo avrebbe dovuto essere opportunità di saggezza per il Governo, che sarebbe potuto intervenire con qualche decreto-legge per modificare le storture o colmare le lacune che ha lasciato indietro. Signora Presidente, se il 5 maggio di questo anno davanti alla Camera e in audizione in Senato si sono dovuti ritrovare gli agricoltori di CIA, Confagricoltura e Copagri per dire, ancora una volta, che la burocrazia soffoca l'agricoltura, significa che, da quand'è iniziato il procedimento (due anni fa), tutto quello che il Governo ha sbandierato come modifiche salutari per l'agricoltura corrisponde a un appesantimento dell'attività burocratica, che è stato quantificato in quattro miliardi di euro all'anno. E, allora, quali sono le benedette riforme di cui vi vantate e di cui il Ministro va nei convegni a prendersi i meriti, che non ci sono?

Questa è anche la difficoltà di concorrenza tra i nostri produttori e quelli europei. E quand'anche ci venisse in soccorso la qualità del nostro prodotto, da troppo tempo stiamo aspettando dal Governo politiche serie in difesa e a tutela del prodotto *made in Italy*. Ricordiamo al Ministro fantasma, che ancora adesso non è presente in Aula, che se qui, quando si è parlato della legge di delegazione europea, non si fossero opposti i Gruppi d'opposizione, Lega in testa, voi avreste approvato una modifica alle nostre normative che voleva cambiare la determinazione del prodotto originario indicando sulla confezione il Paese di ultima trasformazione. Questa era la schifezza che stavate facendo se non ci fossimo opposti noi. E, allora, con che faccia venite a parlare di collegato all'agricoltura come un vantaggio competitivo per i nostri agricoltori? Mi viene da ridere nel leggere quello che diceva il presidente Letta. Diceva che avreste dato ancora più competitività a un settore cruciale, soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi erano strettamente legati all'agricoltura e alla terra. Sempre sarebbe dovuto essere l'anno in cui la preparazione all'Expo e l'agroalimentare italiano avrebbero dovuto produrre la sinergia necessaria al loro reciproco successo. Complimenti! Siete riusciti a chiudere Expo e a passare il semestre europeo senza portare a conclusione questo provvedimento. E ribadisco perché lo sappiano i cittadini che ci ascoltano - che se il Governo vuole, emana decreti-legge che vengono convertiti in legge a Costituzione vigente entro sessanta giorni.

tirare avanti aspettando che la nostra agricoltura sia fatta a pezzi dal CETA o dal TTIP. Mi rivolgo ancora una volta al Ministro dell'agricoltura assente mentre era in giro a tagliare i nastri dei convegni di Coldiretti, il suo collega Calenda era in sede europea a trattare con Juncker per l'approvazione del CETA solo in sede europea, tagliando fuori i Parlamenti nazionali. E, quando noi chiedevamo trasparenza sul TTIP, dov'era il Ministro dell'agricoltura? Su queste cose vogliamo trasparenza e, quando la trasparenza non c'è, significa che l'interesse che sta dietro non è quello dei produttori, non è quello dei cittadini, ma è quello delle *lobby* che hanno a che fare con la finanza, e non con la produzione. Ancora una volta si trasforma l'inganno in beffa, perché i nostri agricoltori non hanno tutela nemmeno rispetto al *made in Italy*. Durante il percorso alla Camera è stato soppresso l'articolo del provvedimento che riguardava la contraffazione alimentare. In quella fase fu detto che era stata insediata la Commissione Caselli, la quale avrebbe dovuto dare entro breve delle linee guida. Il tempo è passato e la Commissione ha concluso il proprio lavoro, che addirittura è diventato oggetto di un disegno di legge da parte del senatore Ruta,

Aspettiamo che l'agricoltura scompaia e, nel frattempo, proiettate anche un bel film per far vedere che vi occupate della tutela della foche monache e saremo anche più contenti e soddisfatti e ci sentiremmo a posto con la coscienza. Vice Ministro, stiamo parlando di agricoltori che tutti i giorni arrivano alla sera senza la certezza di alzarsi il giorno dopo avendo ancora un qualcosa per cui lavorare, la terra. Questo è quanto che sta succedendo. Che cosa non avete fatto su AGEA. L'altro giorno si è dimesso il direttore, ma bastano queste dimissioni per risolvere i problemi di AGEA? Ricordiamo che, nel periodo tra il 15 giugno e l'11 luglio, i nostri agricoltori - non per colpa loro, ma per responsabilità di AGEA - non hanno potuto presentare la documentazione per la PAC e hanno avuto decurtato l'1 per cento al giorno. Di queste cose chi ne risponde? Ne rispondete voi? Ne risponde il Ministro fantasma, che non c'è, che si sottrae anche al confronto?

Non le voglio augurare cattiva salute, per amor del cielo. Vede, Presidente, sono andato a rileggere i Resoconti del 7 maggio 2015 quando in questa sede veniva approvato in prima lettura il provvedimento. Il senatore Ruta, autorevole esponente di maggioranza a cui va tutto il mio rispetto, dichiarava: «Da quanto tempo non si discuteva di un provvedimento così ampio in materia di agricoltura? Certo - lo ricordava poco fa il collega della Lega Nord

ricordando che poi ovviamente ne sarebbero dovuti scaturire provvedimenti di grande attenzione, perché questa mica è una legge, mica è finita qua. Questa è una legge con delega al Governo. Quindi, sappiano gli agricoltori che, una volta approvata in questa sede, il Governo ha tempo ancora dodici mesi e oltre per emanare i decreti attuativi. Quindi, ancora una volta vi dico: fate attenzione agli inganni del Governo perché, quando vogliono, fanno i decreti-legge e sono legge subito; quando a loro non interessano o li usano come spauracchio, diventano provvedimenti che galleggiano per mesi, o anni come in questo caso. Senatrice Bertuzzi - accidenti - ha detto che, per ogni euro di prodotto *made in Italy,* vi sono almeno due prodotti che imitano il prodotto italiano; che 35 sono i miliardi dell'*export* agroalimentare e 60 i miliardi dell'*italian sounding.* Ma che cosa avete fatto per risolvere la questione? Nulla.

e il sistema informatizzato adottato risulta essere di una tale complicazione rispetto alle procedure cartacee adottate fino al 2015 da avere ottenuto un risultato opposto rispetto ai principi di semplificazione. Siamo al paradosso. Avete inserito nuove procedure che, addirittura, complicano la vita

Granieri, ha detto: «Ci voleva più cautela. Ora più controlli nella grande distribuzione». Si stanno infatti accorgendo che le schifezze che vanno sugli scaffali senza neanche la scadenza rischiano addirittura di mettere in crisi la credibilità dell'intero settore.

di procedere velocemente, in modo da concludere il suo esame prima dell'estate 2014. Ma a giugno 2014, semaforo rosso, c'è una coincidenza da aspettare. Era in arrivo il treno (un altro decreto-legge del Governo) dell'alta velocità e della competitività; treno con diversi provvedimenti inerenti il mondo agricolo, che avrebbe assorbito alcuni articoli del collegato. Poi, attraverso accelerazioni e frenate, con date di scadenza di presentazione degli emendamenti continuamente spostate in avanti, siamo giunti alla fine, non senza aver inserito nel collegato numerosi provvedimenti che nulla avevano a che fare con il testo originale. Sono stati aggiunti 8 commi all'articolo 1, e gli articoli 2, 6, 8 , 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Alla Camera hanno soppresso gli articoli 2, 8, 11, 26, 27, 28 e 30 oltre a numerosi commi, per aggiungere gli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 e 41. 40 e 41. E sottolineo l'articolo 38, perché va a correggere l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, la n. 221. Quindi, qui si fanno le leggi e dopo due mesi vengono corrette.

Desidero rimarcare il fatto, peraltro già denunciato, che il Governo prende provvedimenti studiati e analizzati in Commissione, li riassume in pochi commi, li inserisce nel nuovo testo, rendendo pertanto incomprensibile il miglioramento legislativo. In questo provvedimento, che tratta molti argomenti, avete deciso di stralciare l'articolo, molto importante, sulla logistica, elemento di grande importanza per un Paese così lungo e per beni deperibili come le derrate alimentare. I privati investono nel trasporto delle merci, l'*e-commerce* sta crescendo, e voi abbandonate i piani strategici. In questa sede mi limiterò a dire due battute sull'ex articolo 7 del provvedimento del Governo, approvato dal Senato come articolo 9 e che, a seguito dei veri inserimenti, oggi è l'articolo 15. Ricordo che questo articolo era stato riscritto in Commissione al Senato ben sei volte per giungere alla versione definitiva. Pertanto, si potrebbe ritenere che il problema sia stato sviscerato nella sua totalità. Purtroppo, non è così. Alla Camera il testo è stato abbondantemente emendato. È un articolo importante, in quanto delega al Governo la riorganizzazione degli enti partecipati del Ministero delle politiche agricole. Alla Camera è stato aggiunto anche il riassetto del settore ippico, come fosse una quisquilia, una cosuccia da poco. È interessante leggere il comma 2, lettera *e)*: riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol SpA, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero. Come dissi Come dissi un anno fa, sarebbe stato più decente scrivere che il Governo fa quello che vuole. Questo articolo è una delega in bianco a un Governo che non ha idee ed è ancor più sorprendente che, dopo due anni di discussioni, non abbia capito quale sia la risoluzione del problema e non dia una linea di indirizzo precisa. Personalmente la considero un'altra occasione persa: avreste dovuto creare un unico polo dei controlli con il Corpo forestale, ICQRF e Agecontrol, in stretto collegamento con i controlli eseguiti del Ministero della salute. Che il Governo non abbia idee lo si capisce leggendo anche le prime righe di risposta all'interpellanza urgente al Ministro da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera, l'atto 2-00908 dell'anno scorso, sul futuro del rapporto AGEA-SIN. A pochi mesi dallo scadere della convenzione del SIN, non si è ancora arrivati a percorsi normativi per la nuova gara. Vorrei far notare che in Commissione ne abbiamo discusso per un anno e mezzo e sull'argomento le proposte del Movimento 5 Stelle sono precise

Vorrei commentare la situazione attuale di AGEA, per sottolineare quanto sia cronico il disservizio e stigmatizzare l'incapacità del Ministero a metterci una pezza. Già «Il Fatto Quotidiano» del 13 aprile 2015 riferisce Commissione europea ha proposto una rettifica finanziaria per le gravi carenze contestate ad AGEA. In data 24 febbraio 2016 la Commissione europea ha inviato una raccomandata (la n. 956766 del 2016) dove appone delle correzioni negative (sanzioni) ai trasferimenti di fondi all'Italia pari a 158.738.428,33 euro: il fatto che tali debiti non siano stati affatto registrati contribuisce ulteriormente all'asserzione della DG AGRI circa l'esistenza di gravi negligenze nella gestione e nella registrazione dei debiti e di irregolarità da parte dell'organismo pagatore AGEA. Pare altresì che ci sia una lettera di contestazione nella quale Bruxelles avrebbe segnalato 55.000 pratiche relative a finanziamenti stanziati ad agricoltori che non ne avevano diritto, e che la cosa ci costerà 540 milioni di euro. Vice Ministro, risponde al vero l'esistenza di un documento interno ad AGEA nel quale sono state riassunte tutte le rettifiche finanziarie distinte per decisione imputate all'Italia dall'esercizio finanziario 1999 al 2015 per un importo scandaloso di 2.381.319.130,43, che sarebbe il documento che mi è arrivato? Parliamo di trattenute compensate dall'erario per errori, atti falsi, mancati controlli commessi da AGEA, con l'omertà del Ministro delle politiche agricole. Faccio notare che in queste cifre non sono comprese le multe quote latte; anzi, laddove vi è la voce quote latte, sono correzioni positive (quindi soldi che lo Stato italiano ha incamerato). Dai dati in mio possesso emerge, inoltre, che gli scostamenti sono in continuo aumento, soprattutto negli ultimi due anni, evidenziando come la *governance* della struttura non sia all'altezza della situazione: *governance* e dirigenza non brillano per trasparenza e capacità. Rammentiamo che tre funzionari di AGEA, per questi fatti, rischiano il processo in quanto, secondo la tesi della procura, gli indagati «nell'esercizio delle loro funzioni trasmettevano alla Commissione europea le dichiarazioni di affidabilità relative ai conti annuali degli organismi pagatori, omettendo di informare la stessa Commissione del numero effettivo e della reale entità delle posizioni debitorie conseguenti alle erogazioni indebitamente erogate nonché allegando a tali dichiarazioni le certificazioni sulla base di dati da loro stessi forniti e non veritieri». I reati contestati per questi fatti sono abuso d'ufficio e falso; reati a rischio di prescrizione per la legge, ma riferiti a fatti commessi. Approfitto dell'occasione per chiedere la risposta alla domanda che ho posto nel *question time* del 12 febbraio 2015. Nella sentenza T-661 del 2011, subparagrafo 135 viene chiaramente ribadito che l'Italia non ha fatto i controlli e «non possono determinare oggettivamente detto quantitativo». Per questo l'Italia è stata multata per 70 milioni di euro e il Ministro non mi ha mai risposto chi li deve pagare: le Regioni, che non hanno fatto i controlli, o sono soldi che vengono sottratti agli allevatori? Vice Ministro, già nel corso della precedente discussione, avevo lungamente e puntigliosamente evidenziato le incongruità sulla gestione dell'ultima annata delle quote latte 2014-2015. Avevo dimostrato matematicamente come in Italia non ci sono vacche a sufficienza per produrre il quantitativo di latte assegnatoci dall'Europa, il tutto partendo da dati certificati. Avevo anche sollevato l'incongruità di far pagare tanto a pochi allevatori, anziché poco a tutti coloro che avevano superato la loro quota in maniera proporzionata alla presunta superproduzione. Avevo utilizzato parole pesanti contro il fatto che il decreto-legge n. 51 del 2015 cambiava le regole in corsa, scatenando le vostre critiche. Mi ero lamentato perché facevate la cresta, come i bambini: per pagare la multa di 30 milioni di euro, avete preteso il pagamento di 100 Non ho mai capito se i 70 milioni di differenza sarebbero entrati nel fondo latte, per sostenere le aziende in difficoltà che ne hanno pagati 100 - consentitemelo, questo è geniale - oppure se sarebbero serviti per pagare i 70 milioni di multa per i mancati controlli che ho nominato prima. Il 25 maggio 2016 è stata pubblicata la sentenza del TAR di Parma n. 184, che annulla la comunicazione di AGEA per due motivi. Il primo: eccesso di potere sotto diversi profili, per irragionevolezza della imposizione e della normativa di riferimento, anche in relazione alla mancata previa comunicazione della Commissione; secondo: analoghi vizi in relazione alla mancanza di qualsiasi controllo della produzione, come imposto dalle norme comunitarie. Ma sono altre due considerazioni presenti nella sentenza del TAR che meritano un'attenta riflessione: «Con ordinanza collegiale n. 100 del 2016, anche a fronte della incompletezza della difesa erariale (che faceva evidente riferimento ad altra tipologia di controversia)». Sì, avete capito bene: AGEA si è difesa in modo incompleto, presentando al TAR materiare riferito ad altra controversia e - udite, udite - «una memoria ed una relazione tardivamente depositate». E tutti sanno che gli atti presentati in ritardo al TAR sono nulli. Un altro passaggio della sentenza è veramente importante: «assume rilievo dirimente altresì l'ulteriore argomento che contesta il mutamento dei criteri e delle regole di compensazione a campagna chiusa». chiusa». Non sono uomo di diritto, ma un patologo, e c'è soddisfazione nel vedere che le mie considerazioni, dettate dal solo buon senso, sono state condivise da un tribunale. Coloro che hanno scritto e votato siffatto decreto avranno un sussulto di coscienza? Interessante è notare come il nuovo articolo 14 va a correggere l'articolo 2 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, cioé di sei mesi prima;

dell'economia e delle finanze, con oggetto «Criteri di ripartizione e di utilizzazione delle riserve del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 9, comma del 28 marzo 2003, n. 49», si riferisce la nota del dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 37294 del 21 aprile 2016, in cui si sconfessa l'interpretazione del MIPAAF circa l'implementazione del fondo chiedendo la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1. Ho cercato in queste poche battute di evidenziare come una Agenzia così importante per il funzionamento-finanziamento dell'agricoltura, che ripartisce ben 7 miliardi all'anno di fondi europei (PAC), sia allo sbando, e non ho parlato dei ritardi nei pagamenti per non infierire, come ha fatto prima il collega Candiani. Ma quel che è peggio è che, nonostante la cosa sia conosciuta da anni, il Governo non interviene, blocca l'attività del Parlamento con decreti e collegati, ignorando le grida di dolore dei comparti lattiero caseario e suinicolo,

a quelle, assai rilevanti, contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014. In particolare ricordo a me stesso l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole, che è stato un successo e non un accidente della storia o qualcosa che è capitato per caso. Si è trattato di un risultato sicuro e importante, per i possessori di uliveti e per quanti avevano obblighi in materia di prevenzione antincendio e di attribuzione del diritto di prelazione per gli imprenditori agricoli. Si continua a fare semplificazione in materia di costituzione di consorzi di tutela per i prodotti agroalimentari e i vini DOP e IGP,

disposizioni in materia di servitù, stabilendo che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni di gas e per la trasmissione di energia geotermica, per consentire l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali. poi la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. C'è la delega al Governo per il riordino e la semplificazione, attraverso la raccolta delle norme in un codice unico agricolo eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. Pensate che selva di norme esiste in Italia per un agricoltore! Dunque, avere un testo unico in agricoltura è un'esigenza

Il tempo perso nel passaggio tra Senato e Camera è stato esageratamente lungo, ma l'articolo 6 delega il Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante la predisposizione di norme sulle forme dell'affiancamento tra anziani agricoltori o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli; al fine di prevedere criteri di assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali per favorire il processo, definire modalità di conclusione, nonché per stabilire le forme di compartecipazione agli utili proprio delle società di affiancamento per le terre agricole.

per la gestione dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi ad agricoltura e acquacoltura biologiche. Vi sono disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti; all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato si dispone che, qualora sia affidata a terzi, possa essere esercitata esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali in forma cooperativa.

con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e aziende agricole accessibili sul sito Internet di ISMEA per gli utenti registrati. Vengono fornite informazioni su caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei terreni, sulle procedure di accesso alle agevolazioni, sugli eventuali programmi e progetti di ricomposizione fondiaria presentati da ISMEA.

nelle società operanti nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ma anche con interventi a condizioni agevolate attraverso l'erogazione di mutui.

e determinazione. Sul consumo del suolo ci vuole più coraggio e più determinazione nelle scelte, perché stiamo devastando il territorio nazionale e continuando a mangiare terreno per l'agricoltura. Se facciamo lo stesso con la contraffazione, con l'*italian sounding* e soprattutto con quelli che producono cose che proprio italiane non sono, difendendo l'agricoltura italiana e chi trasforma prodotti italiani, rendendo un servizio eccellente al *made in Italy* (quello di cui il mondo ha fame),

aver ascoltato il relatore e i colleghi in questo dibattito, emerge un dato un un dato un po' contraddittorio. Da una parte è stato messo in evidenza l'*iter* legislativo alquanto complesso e in ordine di tempo assai lungo.

che fu fatto un buon lavoro; io allora votai ostinatamente contro, per le ragioni che avevo declinato in quell'occasione.

alla Camera - lo dico soprattutto per coloro i quali non seguono i lavori del comparto agricolo quel testo è stato stravolto. E quando ritornò nella Commissione di merito in Senato, ebbi a sostenere che non era più

di iniziare una serie di audizioni, per meglio capire ed approfondire argomenti totalmente nuovi rispetto al testo precedente. È chiaro che c'è il massimo rispetto per il lavoro fatto dai colleghi deputati, ma il testo comunque rimane completamente stravolto. Per darvi contezza dal testo precedente sono stati soppressi dieci articoli,

siano avvenuti fatti eclatanti nel mondo agricolo, assolutamente no; anzi la richiesta - vero è, per i colleghi che sono intervenuti prima di me - era

indennità espropriative giacenti presso le tesorerie provinciali per mancanza di comunicazione agli espropriati. Sostanzialmente questo articolo, condiviso dal Governo e dalla maggioranza, dà la possibilità di delegare le

sollecitare e intervenire e, ove queste somme non siano per qualche ragione disponibili (nel senso che qualcuno non si è presentato),

la cortesia di occuparci delle somme giacenti nelle tesorerie provinciali? Ma che modo è questo? Certo, presentarsi in un'assemblea di un'organizzazione professionale a enunciare qualche qualche concessione - mettiamola così - e ricevere l'applauso è una cosa che fa piacere a tutti (lo farei anche io). Poi, però, concretamente non vi è nulla dentro quella dichiarazione. Per non parlare - poi - degli enti vigilati. Si tratta di una battaglia che abbiamo fatto in Commissione e in quest'Assemblea. Diteci che cosa volete fare di questi enti vigilati. Siete passati dalla riduzione al riordino, che ci sta bene. ci sta bene. al riordino attraverso le competenze.

Avete soppresso nel Titolo IV

con un confronto leale e vero. Nessuno ci può imporre tempi e corse. Con questo provvedimento, che è per me l'atto più importante per l'agricoltura italiana,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento un anno fa aveva perso per strada molti dei suoi punti qualificanti che erano stati trasferiti in altre misure, ad iniziare dalla legge sulla competitività. Durante la prima lettura avevo sottolineato come questo progressivo svuotamento avesse fatto perdere al provvedimento organicità e impatto. Per questo ho condiviso con i colleghi della Camera l'opportunità di introdurre tutta una serie di modifiche che hanno ridato slancio alla misura, in particolare sul terreno della semplificazione burocratica e dell'attenzione per i piccoli comparti che, a mio avviso, meritano grande attenzione, anche per la funzione di tutela della biodiversità e di utile integrazione al reddito aziendale. Il testo che stiamo discutendo offre un quadro più completo che non si limita alle colture tradizionali, ma interviene anche sui settori che hanno preziose ricadute sul fronte ambientale, sociale e culturale. Penso all'articolo 5, con l'inclusione della silvicoltura e delle filiere forestali nella delega al Governo per un decreto legislativo di semplificazione della normativa. Penso al nuovo articolo 6, che pone l'accento sul tema del ricambio generazionale e dell'ingresso di quelle giovani generazioni che oggi guardano con rinnovata attenzione a un settore nel quale possono portare non solo competenze specialistiche per il miglioramento e l'innalzamento qualitativo della produzione, ma anche saperi e competenze per veicolare nuovi e più salubri stili di vita e di consumo alimentare. Penso alle novità introdotte all'articolo 15 sul riordino degli enti e delle agenzie, che devono essere ripensate per offrire migliori servizi e superare quella pratica odiosa dello stesso controllo effettuato più volte da soggetti diversi, con relativo dispendio di risorse e di tempo sia da parte delle aziende che dello Stato. E, sempre all'articolo 15, la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici, con fonti di autofinanziamento delle associazioni riconosciute, in particolare di quelle delle razze autoctone di montagna, il tutto con l'obiettivo del miglioramento genetico, ma anche della salvaguardia della biodiversità. Importante è anche l'inclusione, all'articolo 21, dei danni causati dalla fauna selvatica tra le compensazioni previste agli agricoltori, assieme a quelle derivanti dalle avversità atmosferiche, dalle epizoozie, dalle fitopatie. Ma apprezziamo altresì il comma 2 dell'articolo 12, con cui si conferiscono alle Regioni e alle Province autonome le modalità di disciplina per i corsi di formazione e per i relativi attestati di idoneità per quei soggetti terzi cui può essere affidata la manutenzione e la sistemazione del verde pubblico e privato. Da ultimo, condividiamo tutte le norme introdotte con gli articoli 33, 34, 35 e 36, che riguardano la produzione di burro, l'apicoltura, le birre artigianali e la produzione del luppolo: settori minori, se ci limitiamo al volume delle produzioni, ma che contribuiscono ad innalzare la qualità e a rafforzare l'immagine della nostra offerta agricola, anche sotto il profilo turistico. In Trentino sono ormai una ventina le aziende che producono birra artigianale, con prodotti di assoluta qualità, un festival dedicato a diversi giovani che, in questo modo, stanno vivendo una importante esperienza dal punto di vista lavorativo o piccolo imprenditoriale. finestra") **(ore 18,51)** (*Segue* PANIZZA). Quindi è un settore da guardare con interesse, anche perché, come sappiamo, ci sono alle spalle anche studi e, in alcuni casi, un'operazione di recupero di antiche tradizioni sulla fermentazione. In questo senso, anche la coltivazione del luppolo può costituire una possibilità per il recupero di tutta una serie di terreni incolti o abbandonati, soprattutto nei territori di alta montagna. Ma questo del luppolo è solo un esempio delle attenzioni che meritano le piccole realtà, dove deve essere sempre più favorito l'approccio plurifunzionale. Strategico è a questo punto il settore dell'agriturismo, perché offre un'esperienza emotiva al turiste e all'ospite, perché rafforza il senso di identità e di appartenenza a una comunità, ma anche perché contribuisce, quando poi i turisti e i clienti tornano a casa, a riproporre e consumare ancora i prodotti che hanno conosciuto sul territorio, insieme alla loro esperienza di produzione e la cultura che esprimono. In quest'Aula e in Commissione ho parlato diverse volte dell'importanza dell'agricoltura di montagna come antidoto allo spopolamento, come strumento per la salvaguardia della biodiversità, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la piena valorizzazione del patrimonio etnografico, naturalistico e paesaggistico montano. L'agricoltura di montagna è fondamentale per la coesione sociale, per la vitalità di un territorio, per il suo sviluppo turistico, per la possibilità, attraverso la specificità delle produzioni, di conferirne una forte riconoscibilità in termini dì *marketing*. Attendiamo, al riguardo, le norme attuative del provvedimento sull'agricoltura sociale. Ma soprattutto crediamo che tutte le politiche per l'agricoltura di montagna debbano aiutare le imprese a fare reddito, abbattendo i costi, semplificando la burocrazia, favorendo sempre più l'accesso dei giovani, anche con modalità *part-time*, perché se non guadagnano e non possono investire le aziende purtroppo muoiono e i giovani se ne vanno. La semplificazione burocratica deve restare uno dei punti focali di tutti i nostri interventi legislativi, ad iniziare dai futuri decreti legislativi legati agli articoli 5, 6 e 15 di questo provvedimento. Non dimentichiamolo, ogni volta che introduciamo una nuova norma, anche quando questa è mossa dalle migliori intenzioni, per le piccole aziende si traduce in un carico di burocrazia e di adempimenti che portano via tempo e risorse al lavoro e alla produzione o, peggio ancora, non sono di sostegno alle aziende. Voglio fare anche un accenno alla regolamentazione dei pesticidi, un tema che si sta sempre più rivelando di grande importanza. Io credo che occorra operare con grande attenzione, perché è assolutamente necessario ridurne l'uso, sia perché il mercato va giustamente nella direzione di prodotti che rispettano determinati *standard* durante la coltivazione, sia per tutelare la salute del consumatore, ma anche dei coltivatori, a causa delle prolungata esposizione a tali prodotti. Ma non dimentichiamoci che, in alcuni casi specifici, vi è anche un tema di costi, che in qualche modo devono essere compensati se vogliamo che l'utilizzo dei pesticidi sia ridotto allo stretto necessario. Tuttavia, ci possono essere delle situazioni nelle quali bisogna farvi ricorso per l'eliminazione dei parassiti e la salvaguardia del raccolto. Sui piccoli frutti viviamo in queste settimane in Trentino la rapida e pericolosa diffusione della *drosophila suzukii*, un moscerino che, per le basse temperature e l'elevato tasso d'umidità, sta trovando il clima ideale per la sua diffusione. I trattamenti fitosanitari consentiti non sono in grado di risolvere il problema, mentre l'utilizzo fino agli anni scorsi di altri prodotti autorizzati in via eccezionale permettevano il controllo dell'insetto. È solo un esempio, ma rende bene l'idea della necessità di aprire delle finestre temporali, del tutto eccezionali e legate a situazioni specifiche, in cui si deve consentire l'uso di prodotti che possono salvare i raccolti senza comprometterne la salubrità. È poi giunto il momento di una riforma radicale nel settore della ricerca. In questi anni si è speso molto, con risultati non sempre all'altezza delle risorse impiegate. Bisogna mettere in collegamento le varie strutture, puntando all'efficacia e ai risultati. Dobbiamo, in una parola sola, fare sistema. Così come diviene sempre più importante la lotta alla contraffazione del nostro agroalimentare, che costituisce un danno ingentissimo per le aziende, per l'erario, per l'immagine del nostro Paese e dei nostri territori. L'Europa, anche in questo settore, continua ad apparire come un'istituzione vessatoria, con i suoi continui *Diktat* burocratici, ma, soprattutto, distante dai problemi e dai bisogni del settore. Pensiamo all'abolizione delle quote latte, ma pensiamo anche all'ipotesi su cui si era ragionato a Bruxelles, fortunatamente scongiurata, di liberalizzare l'utilizzo dei nomi dei vini che avrebbe aperto un'autostrada alla contraffazione dei nostri marchi più pregiati. Un tema, quello della lotta alla contraffazione e sulla rintracciabilità della storia del prodotto, sul quale si sono spese molto le organizzazioni professionali, anche con significative manifestazioni, come quelle sul Brennero, su cui anche l'Europa deve essere più solerte nel dare risposte al nostro Paese. Su tutti questi temi, come autonomisti trentini, abbiamo presentato un documento programmatico al Ministro, con tutta una serie di proposte concrete per la semplificazione burocratica e la valorizzazione del settore. Perché l'agenda delle priorità è molto lunga, e non viene di certo esaurita con questo provvedimento o con quelli, seppur importanti, che da inizio legislatura sono stati approvati. Per tornare al collegato, adesso che finalmente siamo in dirittura d'arrivo anche in un testo completamente stravolto rispetto a quello iniziale, io credo gli vadano riconosciuti due meriti. Il primo è di aver posto, a inizio legislatura, il tema agricolo come uno dei temi strategici per il rilancio della nostra economia, aiutandolo ad uscire da quella marginalità in cui a un certo punto era caduto. Il secondo è quello d'aver recuperato, con un colpo di reni, una visione d'insieme anche sugli aspetti sociali, ambientali, direi anche culturali, del settore. Doveroso, alla fine di questo lungo percorso, un ringraziamento al relatore, senatore Formigoni, ai componenti della 9a Commissione, ai rappresentanti del Governo, in particolare al vice ministro Olivero, che ha seguito tutto l'*iter* del provvedimento alle organizzazioni professionali, per lo spirito collaborativo che ha sempre animato le nostre discussioni e nostri lavori. Spirito che, ne sono certo, manterremo anche nei prossimi provvedimenti che ci aspettano, e che sono di grande importanza, se davvero vogliamo che questa legislatura lasci un segno tangibile e concreto sul comparto.

vorrei innanzitutto sottolineare che le disposizioni del disegno di legge oggi in discussione sono molto importanti, perché danno risposte concrete ed intervengono su molti aspetti di rilievo del settore agricolo, introducendo significativi cambiamenti, semplificazioni ed innovazioni. Penso all'articolo 6, che disciplina le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantenni o pensionati e i giovani, al fine di incentivare quel ricambio generazionale di cui l'agricoltura ha molto bisogno per accrescere il suo potenziale competitivo. Una disposizione che risulta ancor più importante ed urgente, alla luce del rapporto ISTAT sullo stato di salute dell'agricoltura italiana, dal quale emergono le criticità ed il persistere di gravi problemi che attanagliano la nostra agricoltura. Ne cito solo due, quelli che, a mio parere rappresentano le due principali criticità, strettamente correlate fra loro. Da un lato, il fatto che il valore dei prodotti finisce in grandissima parte all'industria della trasformazione e alla distribuzione; dall'altro, la continua diminuzione, in termini numerici, dei giovani agricoltori. Occorre, quindi, mettere in campo ogni iniziativa rivolta a favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura e la misura prevista in questo provvedimento va in questa direzione. Penso poi all'introduzione della Banca delle terre agricole, presso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per meglio coordinare il percorso già avviato a livello regionale, come, ad esempio, in Emilia-Romagna, dove è stato presentato uno specifico progetto di legge al riguardo, rivolto all'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate a fini produttivi. Ritengo poi molto rilevante la semplificazione introdotta per le reti di impresa costituite nella forma di reti contratto; una semplificazione che potrà incentivare le nostre imprese ad organizzarsi insieme, favorendo in questo modo sinergie per innovare e competere. Finora sono stati stipulati 2.500 contratti: più di 400 di questi riguardano proprio il settore agroalimentare, con quasi 1.500 imprese coinvolte, nel settore del latte, nell'ortofrutticoltura, nell'agricoltura di precisione, nell'agriturismo. Sono pratiche positive che, grazie alle semplificazioni introdotte con questo provvedimento, potranno essere estese e allargate. Molto importante è la risposta data ad alcune filiere, come l'ippica, che si trova in una situazione di gravissima difficoltà. Con la delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale, l'Esecutivo è impegnato ad attivarsi con urgenza per garantire una nuova forma di *governance* in grado di rilanciare un settore che nel nostro Paese può contare, oltre che su una grande tradizione, su un ingente patrimonio di razze, di competenze, di strutture dedicate. A proposito di nuove filiere, vorrei sottolineare la positività dell'intervento che tende ad accompagnare la crescita di una nuova filiera che sta conoscendo una buona espansione commerciale. Mi riferisco alla crescita - non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi dei birrifici italiani che producono birra con metodo artigianale. Con il collegato si colma una lacuna legislativa, introducendo una definizione che permetterà l'assegnazione dell'attributo di birra artigianale, indispensabile per la piena valorizzazione Va in questa direzione anche l'intervento per favorire, con uno specifico finanziamento, la coltivazione della materia prima, con l'avvio di progetti di ricerca per la produzione del luppolo e la ricostituzione del relativo patrimonio genetico. Molto positivo è il sostegno alla filiera corta e al biologico, un modo di fare agricoltura che coniuga sostenibilità ambientale, salubrità, valore del lavoro agricolo. Voglio infine citare una norma che introduce, nell'ambito della rappresentanza nei consorzi di tutela, per gli amministratori di questi consorzi, il principio dell'equilibrio tra ì generi. Si avvia, quindi, anche in questo ambito di rappresentanza un percorso graduale che, tenendo conto della natura e delle peculiarità delle rappresentanze associative, potrà assicurare un apporto significativo e - ne sono convinta - di valore da parte delle donne oggi ancora sottorappresentate. un'ultima e generale considerazione. In questa legislatura è stata dedicata, come occorreva, grande attenzione all'agricoltura, quella attenzione che meritava da tempo. Voglio ricordare, in estrema sintesi, alcuni provvedimenti che abbiamo avuto modo di esaminare e approvare in quest'Assemblea: dal decreto-legge competitività al rilancio dei settori in crisi, al tema della riorganizzazione degli enti e delle relazioni all'interno delle filiere. Sono state, poi, molto importanti le norme contenute nell'ultima legge di stabilità: l'eliminazione di IRAP e IMU sui terreni agricoli. Di questa mole di interventi va dato merito al Governo, al ministro Martina, al vice ministro Olivero, oltre che al lavoro delle colleghe e dei colleghi della Commissione agricoltura. La grande attenzione al settore agricolo in questa legislatura ha promosso rilevanti interventi per favorirne la crescita in termini quantitativi e qualitativi, e per dare risposte importanti anche in ambito sociale. Ricordo a questo proposito il disegno di legge approvato sull'agricoltura sociale. L'agricoltura è un settore sul quale puntare con decisione, ha una grande potenzialità di crescita e costituisce un imprescindibile elemento per lo sviluppo dei nostri territori. Può rappresentare - e i recenti dati sull'aumento dell'occupazione nel settore lo confermano, così come i dati sul valore sull'*export* agroalimentare - un settore strategico per accrescere l'occupazione, in particolare giovanile. Per questo occorre fornire strumenti adeguati e migliorarli: formazione, accesso alla terra e al credito. Per questo occorre utilizzare al meglio nei territori i programmi di sviluppo rurali, che hanno misure per favorire l'insediamento dei giovani. Dobbiamo infine sempre ricordare che l'agricoltura costituisce un presidio indispensabile per la manutenzione e la salvaguardia del territorio, quel territorio che è espressione del valore culturale, paesaggistico ed ambientale del nostro Paese; un territorio agricolo, nel quale si sta sviluppando un'offerta di turismo importante che punta sempre più sul binomio paesaggio ed enogastronomia, che sono il segno distintivo di una buona agricoltura. Una buona agricoltura, che con questo provvedimento vogliamo incentivare ed aiutare, con un pacchetto di misure che hanno obiettivi molto concreti: semplificare, innovare, riorganizzare, sostenere. Interventi necessari per affrontare meglio le enormi sfide ed i problemi legati alla competitività internazionale, che mette in difficoltà le nostre imprese, che per questo motivo vanno sempre più e meglio sostenute. Signor Presidente, arriva oggi al termine del suo *iter* un provvedimento che è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria del 2014; percorso che, proprio in ragione del lungo periodo trascorso, avrebbe dovuto avere la possibilità di mettere in campo misure in grado davvero di rilanciare l'agricoltura. Il comparto agricolo del nostro Paese affronta quello che doveva essere un anno decisivo per il suo sviluppo, con il traino di quello che avrebbe dovuto essere l'Expo di Milano, in un quadro però fortemente compromesso dalle troppe crisi di settore e dall'assenza di un chiaro indirizzo di politica agricola nazionale, con gravi ripercussioni sulla sua redditività. Le grandi potenzialità del prodotto agricolo e agroalimentare italiano nel mondo sono di fatto limitate fortemente proprio dall'incapacità politica, ormai decennale, di esprimere orientamenti chiari a sostegno dei settori strategici che soffrono, con sempre maggiore evidenza, la concorrenza internazionale. Sono in forte difficoltà alcuni comparti decisivi per il modello alimentare del nostro Paese. In crescente sofferenza sono le aziende ortofrutticole, esposte al dinamismo delle esportazioni spagnole e nordafricane; il settore del latte e dell'allevamento bovino, con una drastica riduzione delle aziende attive; il comparto cerealicolo, che vede ridursi progressivamente il contributo della produzione nazionale; il settore olivicolo, anche per effetto della fitopatologia che sta interessando la Puglia, alla quale, anche in questo provvedimento, non si è voluto dare una risposta efficace. Inviterei su questo il Ministro e i rappresentanti del Governo ad un'adeguata riflessione critica, perché non è più tollerabile sottovalutare ancora questa emergenza per l'agricoltura e l'ambiente, che rischia di sconvolgere per sempre un paesaggio, un'economia e una coltura strutturale per gran parte del nostro Paese. Difficoltà che certamente hanno origine dalla crescente concorrenza internazionale, ma anche da ragioni più specificamente legate alle condizioni strutturali del settore nel nostro Paese. Mi riferisco in particolare al perdurante divario che sussiste fra una produzione agricola fortemente frammentata, dove prevale tuttora la piccola azienda familiare, ed una distribuzione ben più fortemente organizzata, dove ormai cinque grandi piattaforme - cinque! determinano oltre il 70 per cento degli acquisti alimentari, con le conseguenze evidenti in termini di squilibrio dei poteri. In pratica, il valore aggiunto della produzione tende costantemente a trasferirsi dalla produzione alla distribuzione, con gli agricoltori che si trovano ormai a fronteggiare margini di redditività sempre più ristretti, insufficienti e, in alcuni casi - mi riferisco in particolare al settore del latte - inesistenti. Per fronteggiare la crisi e ridare slancio all'economia agricola occorrono un indirizzo e un progetto chiaro che, obiettivamente, non riusciamo proprio a rintracciare in questo provvedimento, che potremmo definire senza infamia e senza lode. Il disegno di legge collegato agricolo era nato con altre ambizioni - almeno così avevate detto, colleghi della maggioranza - mentre il contenuto concreto che oggi ci apprestiamo a votare, nonostante alcuni sforzi effettivamente fatti in Commissione, in prima lettura, non presenta quel carattere di organicità che era auspicabile. Siamo di fronte ad un insieme di norme raffazzonate, in alcuni casi confuse, ancora una volta prive di un filo conduttore e di una direzione di marcia univoca. La prima parte del provvedimento presenta alcuni spunti interessanti sulla semplificazione burocratica, che rischiano però di essere vanificati dalle modalità di recepimento decise per la riforma della politica agricola comune, laddove si preannunciano gravi appesantimenti burocratici per gli imprenditori agricoli. Ancora una volta si profila, su questo aspetto decisivo, un'occasione mancata per snellire gli adempimenti amministrativi e fiscali degli agricoltori e il loro rapporto con gli enti pagatori. Certamente più innovativi e interessanti appaiono alcuni elementi introdotti in Commissione e durante l'esame alla Camera dei deputati, quali l'istituzione della Banca delle terre agricole e le nuove disposizioni che definiscono la birra artigianale, un fenomeno in crescita e di sicuro interesse anche per le imprese agricole. Rilevanti sono anche le norme specifiche che riguardano la filiera del pomodoro e del riso. È stato invece soppresso, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il nostro emendamento istitutivo dell'articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica per il comparto agroalimentare. Ci auguriamo che il Governo voglia tornare quanto prima su questa problematica, in quanto la modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso, dei trasporti e delle piattaforme logistiche per l'esportazione dei nostri prodotti è un fattore decisivo, anche per sconfiggere quelle ecomafie, che proprio sull'arretratezza dei trasporti agroalimentari hanno costruito il loro controllo sulle filiere. Abbiamo inoltre proposto, sia in Commissione che in Assemblea, senza incontrare il consenso della maggioranza, un intervento a favore dei Piani di settore, già approvati dal Ministero delle politiche agricole, che interessano filiere di rilievo strategico, senza che si siano prodotti risultati apprezzabili, in assenza di un adeguato fondo di finanziamento. È stata inoltre respinta in Commissione una nostra proposta rivolta ad affrontare la problematica dell'abbandono dell'attività agricola nelle aree interne del Paese, uno dei fenomeni più preoccupanti non solo per la tenuta complessiva del settore, ma, in particolare, per le evidenti conseguenze sull'assetto idrogeologico del Paese, derivanti dall'interruzione delle attività di manutenzione continua del territorio storicamente assicurate dagli agricoltori. I danni da fauna selvatica al settore agricolo, in gran parte riconducibili alla diffusione del cinghiale, continuano ad essere fonte di rischio per il settore e occasione di conflitto fra gli agricoltori e gli enti locali, con particolare riferimento alle aree naturali protette. Anche su questo abbiamo sollecitato e continuiamo a sollecitare un intervento tempestivo del Governo, a fronte delle crescenti difficoltà che vengono segnalate dalle organizzazioni professionali agricole, agricole, che tenga conto della necessità di rafforzare le azioni di prevenzione dei danni. Auspichiamo infine che sia affrontata adeguatamente e con urgenza la questione del caporalato, oggetto attualmente di uno specifico disegno di legge all'esame della Commissione agricoltura, questione sulla quale registriamo complessivamente un ritardo di interpretazione e di intervento, che rischia di farci assistere ad un'altra stagione delle raccolte senza che siano stati predisposti gli strumenti di prevenzione e controllo necessari per sradicare il fenomeno dalle nostre campagne. In conclusione, questo provvedimento che, lo ripeto, appare senza infamia e senza lode, a nostro avviso non è assolutamente in grado di dare risposte efficaci a un settore che, nonostante i gravi problemi, è uno dei pochi che ha tenuto in questa situazione di crisi e che avrebbe avuto bisogno di un'opportunità di rilancio e di intervento. Sollecitiamo quindi il Governo ad aprire ben altri spazi di discussione e di iniziativa a favore dell'agricoltura italiana nell'ambito del decreto-legge già esaminato dal Consiglio dei ministri sulla questione del latte e nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica. Noi di Sinistra Italiana riteniamo anche che sia necessario ribadire con chiarezza la posizione italiana sugli organismi geneticamente modificati e sul loro utilizzo in agricoltura, questione sulla quale registriamo nuovamente nel Governo posizioni equivoche, che possono dare spazio a chi vuole rimettere in discussione un orientamento di precauzione assunto con il pieno consenso del mondo agricolo nazionale. Non mancheremo dunque di incalzare ancora il Governo nella convinzione che le difficoltà del settore agricolo richiedano ben altro supporto, anche finanziario.

l'Assemblea esamina oggi un provvedimento organico per il settore agricolo, che offre risposte concrete ad alcune importanti filiere in difficoltà e accompagna e meglio definisce il processo di innovazione e semplificazione del comparto produttivo primario, avviato fin dall'inizio della legislatura. Questa è, per l'agricoltura italiana, una legislatura storica, caratterizzata da un grande protagonismo del Parlamento e del Governo in favore del settore primario. L'attenzione dedicata a tale comparto nasce dalla consapevolezza che l'agricoltura è un settore con straordinarie potenzialità, ma che, allo stesso tempo, sta attraversando grandi problemi legati a una competitività internazionale sempre più libera e quindi sempre più aggressiva nei confronti delle nostre imprese. È un settore attanagliato da un contesto di burocrazia che in molti casi ne blocca molto la capacità espressiva; è un settore che ha molte complessità e anche molte debolezze legate alla storia che ne ha fin qui caratterizzato il divenire. Il settore agricolo negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nell'economia e nello sviluppo del Paese e ora, anche grazie alle misure contenute nella legge di stabilità per il 2016, ha quasi un miliardo di risorse: una grande occasione per rafforzare e potenziare filiere, accrescendone la qualità mediante coltivazioni sempre più sostenibili e attente all'interesse del consumatore. In questa prospettiva si registra la significativa ripresa del comparto agricolo nazionale, evidenziata soprattutto dall'incremento delle esportazioni agroalimentari. Si tratta di un risultato importante, che premia gli sforzi degli imprenditori agricoltori che hanno saputo resistere alla grande crisi economica, agganciando la ripresa ben prima di altri comparti economico-produttivi: basti solo pensare che nell'ultimo anno il vino italiano ha superato in quantità e in qualità il vino francese. Le principali direttrici che hanno orientato la nostra attività legislativa in tema di agricoltura si possono sintetizzare in poche parole: semplificazione burocratica, riduzione del peso fiscale, accesso al credito, sostegno al lavoro in agricoltura, ricambio generazionale, rafforzamento del tessuto produttivo e competitività. Entrando negli merito del provvedimento, desidero in primo luogo ricordare il proficuo e straordinario lavoro svolto dal Senato in prima lettura. Sono state in tale occasione definite disposizioni estremamente innovative e rilevanti per l'agricoltura: penso all'articolo 6, che disciplina le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantenni o pensionati e i giovani, al fine di incentivare quel ricambio generazionale di cui l'agricoltura ha molto bisogno per accrescere il suo potenziale competitivo. Penso poi all'introduzione della banca delle terre agricole presso l'ISMEA, per meglio coordinare quel processo avviato già in ambito regionale rivolto all'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate a fini produttivi. La Camera ha approvato dei correttivi e degli idonei aggiustamenti dovuti al concatenarsi in questi mesi di provvedimenti legislativi approvati che hanno riguardato direttamente o indirettamente il comparto, al fine di evitare che potessero verificarsi sovrapposizioni, incongruenze o contrasti con altre riforme poste nel frattempo in essere. Per questo, la Camera dei deputati ha ritenuto che la revisione delle norme penali in materia di contraffazioni andasse necessariamente coordinata con il lavoro che ha iniziato a svolgere la commissione di studio per la riforma dei reati agroalimentari, istituita presso il Ministero della giustizia ed ha pertanto soppresso l'articolo 2 del testo licenziato in prima lettura. modo, gli articoli 8 e 11 sono stati soppressi in quanto, intervenendo in materia di subappalto e di logistica nel settore agroalimentare, richiedono necessariamente un coordinamento con la riforma del codice degli appalti da poco approvata. In merito alle disposizioni riguardanti la pesca e l'acquacoltura, è stato necessario mantenere solo le disposizioni relative alle sanzioni per la pesca illegale, avente un carattere di estrema urgenza per risolvere il contenzioso che si è aperto con Bruxelles in merito, per esempio, alla cattura delle vongole (sappiamo che oggi è stato approvato il provvedimento che ha ridotto la taglia a 22 Le altre necessarie disposizioni saranno oggetto di approfondimento e di valutazione nell'ambito dell'esame di un apposito provvedimento sulla filiera ittica, il cui *iter* è già in una fase avanzata presso l'altro ramo del Parlamento. Sono state invece introdotte, in maniera speculare rispetto alla pesca illegale in acque marine, specifiche sanzioni per il bracconaggio nelle acque interne: un tema molto caro alle diverse forze politiche, che ha trovato un punto di storica soluzione. È importante inoltre sottolineare come sia stata inserita una delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale. Il comparto si trova in una situazione di grave difficoltà e, per non disperdere il grande patrimonio di razze e di competenza che caratterizza la filiera, occorre muoversi con urgenza, per assicurare una nuova ed inclusiva forma di *governance*, capace di risollevare e rilanciare il settore. Altro intervento di rilievo è quello che riguarda il settore della birra artigianale, cioè quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. e microfiltrazione. Pensiamo alla straordinaria esperienza di numerosi birrifici italiani (oramai siamo quasi arrivati a novecento), che hanno dapprima sperimentato e poi lanciato sul mercato il nuovo prodotto della birra ottenuta con metodo artigianale. Numerosi piccoli produttori nazionali hanno conseguito in questi ultimi anni un successo straordinario, promuovendo nei fatti anche l'inizio di un movimento come quello alogastronomico, che pare stimolare in modo qualificato anche lo sviluppo turistico. Ad oggi mancava una definizione legislativa che permettesse loro di poter definire l'attributo artigianale: con il collegato abbiamo colmato questa lacuna, ponendo le basi per un'ulteriore ed efficace valorizzazione, che mi auguro possa avvenire al più presto. La produzione della birra, in particolare quella artigianale, soffre poi nel nostro Paese della carenza di materia prima: ogni possibile espansione del settore richiede quindi l'avvio di progetti di ricerca per la produzione del luppolo, anche attraverso la ricostituzione del relativo patrimonio genetico e l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Il collegato, a tal proposito, prevede un finanziamento specifico per la coltivazione del luppolo. Altro tema rilevante, è la necessità del settore apistico di avere un sistema di riconoscimento certo dei prodotti. A tal fine, mentre abbiamo approvato modifiche significative nel comparto dell'apicoltura, abbiamo introdotto alcune semplificazioni e talune sanzioni per coloro che non denunciano la detenzione di alveari all'anagrafe apistica. Abbiamo valorizzato la filiera del riso, anche come espressione del valore culturale, paesaggistico ed ambientale di un territorio, tutelandone le varietà tipiche, garantendo la qualità e la tracciabilità e prevedendo la possibile revisione della normativa istitutiva istitutiva dell'Ente nazionale risi nell'ambito della delega al Governo. Abbiamo inoltre introdotto il principio dell'equilibrio tra i generi anche per gli amministratori dei consorzi di tutela, prevedendo un percorso di graduale approdo che tenga conto della natura e delle peculiarità delle rappresentanze associative, anche in riferimento alla caratura delle espressioni. Infine, abbiamo reso possibile una maggiore trasparenza nel sistema allevatori. Da ultimo, intendo sottolineare una norma non propriamente agricola (mi piace definirla collaterale), che tuttavia ha trovato spazio in questo provvedimento: è la norma che in qualche modo consente agli sfalci, alle potature e alla paglia di poter essere utilizzati non più come rifiuti, ma come risorse per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Ebbene, questa è una norma di straordinaria civiltà, oltre che di sostanza, perché consentirà ai Comuni, ovvero ai cittadini, di risparmiare risorse preziose. Come ho cercato di illustrare, seppur brevemente, si tratta di un provvedimento ricco di contenuti, elaborati e migliorati da entrambi i rami del Parlamento, la cui approvazione darà ulteriore spinta propulsiva ad un settore in costante crescita e verso cui indirizzare l'attenzione nel prossimo futuro per una crescita sostenibile del nostro Paese.

oggi in discussione un provvedimento che, a detta dei proponenti, è stato concepito per rendere il settore agricolo più semplificato e, quindi, più snello, veloce e probabilmente anche più competitivo, ma che, in realtà, non fa altro che renderlo ancora più contorto, complicato e probabilmente anche arcaico. Si pensi soltanto che si va dal dettare disposizioni in materia di produzione della birra artigianale alla denominazione del fungo cardoncello, dal riassetto del settore ippico a numerose deleghe al Governo per il rilancio di alcuni settori chiave e persino all'introduzione della parità tra i sessi nei consorzi di tutela. In occasione dell'approvazione in prima lettura in quest'Aula, ho avuto modo di dichiarare il voto contrario di Forza Italia al disegno di legge originario, successivamente modificato dalla Camera dei deputati. ritenevamo che quel testo fosse poco adatto al rilancio della competitività del settore agricolo, in quanto quasi tutte le disposizioni aumentavano di gran lunga gli oneri burocratici. Oggi come ieri, il mio giudizio non si discosta dal precedente. Si fa fatica a trovare anche una sola disposizione che vada nella direzione di una riqualificazione e semplificazione del settore agricolo.

introdurre nuovi limiti e divieti anziché eliminarli e inserire deleghe su deleghe al Governo anziché semplificare la normativa, è del tutto contraria agli obiettivi che ci si era prefissati. Il settore agricolo e, più in generale, tutti i settori su cui il provvedimento incide, hanno una grande rilevanza per la nostra economia e non dovremmo mai, in alcun modo, disincentivarne lo sviluppo. Si dovrebbe snellire, sburocratizzare, incentivare l'iniziativa imprenditoriale e provvedere a un regime fiscale semplice, snello, giusto e veloce. Il disegno di legge in esame contraddice invece in ogni sua parte le ricette dell'economia liberale, volte a dare sostegno all'iniziativa privata e alla crescita economica. di un'Italia che, con tutte le leggi prodotte, ha soffocato la buona volontà di milioni di cittadini che, con la loro operosità, avrebbero certamente contribuito alla crescita del nostro Paese. Non solo un così alto grado di burocrazia non fa altro che rendere il terreno sempre più fertile per far attecchire e diffondere il malaffare, ma proprio il *referendum* di qualche giorno fa del popolo inglese per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea

è del tutto contraria rispetto all'obiettivo prefissato. Il settore agricolo e, più in generale, tutti i settori su cui il provvedimento incide hanno una grande rilevanza per la nostra economia e non dovremmo in alcun modo disincentivarne lo sviluppo. Si dovrebbe snellire, sburocratizzare e incentivare l'iniziativa imprenditoriale e si dovrebbe, pertanto, provvedere a un regime fiscale semplice e giusto. Il disegno di legge in esame contraddice invece in ogni sua parte le ricette dell'economia liberale, e fa della burocrazia il principale nutrimento proprio per complicare la strutturazione dei provvedimenti. Del resto, gli inglesi hanno manifestato, a ragione, la volontà di opporsi a ciò che in concreto produce l'Europa: regolamenti dettagliati, cavilli burocratici sui millimetri delle vongole, regole economiche che non tengono conto degli equilibri in *surplus* della Germania e, poi, fiumi di chiacchiere in occasione dei Consigli europei. Delle grandi sfide che necessitano di interventi urgenti e mirati, come la grande crisi migratoria, nemmeno l'ombra. È sicuramente un avvenimento di portata storica, ma, dal punto di vista politico, la Brexit deve darci uno spunto di riflessione. Occorre ripensare, con grande umiltà, che costruendo torri d'avorio, così separate dalla vita dei cittadini, così distanti dal prendere in considerazione le voci di cambiamento, così rigide di fronte ai problemi economici e sociali, si rischia spesso di vederle crollare. Un monito va anche a questo Governo che, con questo e simili provvedimenti, va nella direzione sbagliata. Non semplifica, non riordina e non innova in maniera adeguata il settore agricolo; anzi, lo rende ancora più saturo di adempimenti e oneri burocratici e ciò sicuramente non si tradurrà in competitività del settore agricolo, che è invece un settore trainante per l'economia e per il PIL italiano.

tra le due Camere, ma è anche vero che affronta temi fondamentali del settore agricolo. Fin dall'inizio abbiamo considerato questo testo una sorta di legge quadro per la complessità dei temi fondanti che affrontava. Nel corso di questi due anni le modifiche sono avvenute per ulteriori approfondimenti fatti alla Camera perché, in parallelo, alcune misure si sono concretamente attuate. inseriti nuovi temi, come il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico con maggiore coordinamento e controllo da parte del Ministero o come quello, determinante, dell'apicoltura. Vista l'importanza di questo settore e i rischi fitosanitari che affronta costantemente, viene previsto un più stretto controllo e rigore con l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia delle variazioni di alveari all'anagrafe apistica nazionale. Su questo voglio esprimere soddisfazione per un ordine del giorno che ho presentato e che è stato accolto, del quale il Governo ha condiviso la preoccupazione espressa dalle organizzazioni apistiche perché ci sia un uso puntuale, rigoroso e non generalizzato della sanzione,

Il settore apistico è nei fatti e non nelle opinioni precondizione dell'intero ciclo vegetale. Senza le api non c'è impollinazione e, quindi, niente biodiversità, niente piante e, quindi, niente animali. Non abbiamo abbastanza presente questo. È un settore fondamentale e le minacce di parassiti devastanti da qualche anno stanno fortemente preoccupando produttori e istituzioni. La mia Regione, la Liguria, sta vivendo in modo drammatico parassiti come la vespa vellutina, il calabrone asiatico e l'aethina tumida, che viene citata proprio in questo provvedimento. Più volte ho portato all'attenzione della Commissione e dell'Assemblea questo tema. L'aethina tumida è un parassita che si nutre dei favi, della cera e di tutto ciò che trova nella casa delle api. Il miele contaminato diventa inutilizzabile mentre l'arnia, distrutta, è colonizzata dalle larve. Il parassita può deporre fino a 2.000 uova. Se non si tiene un controllo rigoroso, l'intero mondo dell'impollinazione può essere compromesso con conseguenze devastanti. Dico questo perché, al di là dell'articolo specifico dedicato all'interno del collegato agricolo, è evidente come la questione della prevenzione, di un sistema fitosanitario nazionale e territoriale rafforzato e maggiormente collegato al sistema della ricerca sia un tema fortemente prioritario. I nostri valori ambientali più pregiati sono a forte rischio se non riusciamo ad adeguare strumenti di forte contrasto e conoscenza delle minacce nuove che arrivano. Parlo delle api come degli ulivi con la *xylella* o dei castagneti di tutta Italia con l'infestazione della vespa cinese, fino all'ultima arrivata: la cimice asiatica, che sta minacciando seriamente i frutteti dell'area bolognese e a proposito della quale il collega Broglia si sta facendo, proprio in questi giorni, interprete delle preoccupazioni dei produttori. E potrei parlare di decine e decine di esempi preoccupanti. Un provvedimento come il disegno di legge n. 1328, che affronta i temi fondanti della crescita di competitività, non può dunque che partire dalla tutela della salute delle proprie produzioni; deve introdurre una nuova impostazione della gestione della mobilità globale dei parassiti, una gestione strutturata e rapida nel

Alcune deleghe, come quella per il settore della pesca, sono state stralciate per impostare un provvedimento dedicato, che è già in corso di approvazione alla Camera. Sono invece rimaste le disposizioni relative alla pesca illegale, modificate ed adeguate al sistema sanzionatorio delle disposizioni europee. Sono state inserite sanzioni per il bracconaggio nelle acque interne. Il provvedimento in discussione contiene, secondo me in modo utile, una dimensione generale di riforma e di semplificazione di leggi, sovrapposizioni di leggi, procedure e strumenti di gestione pubblica mi riferisco alla riforma degli enti, che è già in corso - ma affronta anche la gestione dei singoli comparti che hanno esigenza di percorsi di valorizzazione, di una di una qualità certificata e garantita da una seria tracciabilità, quei settori che sono maggiormente esposti ad una competizione globale, in onde di ingresso difficilmente sfidabili se non sui livelli di identificazione e di alta qualità e trasparenza. Questo, sia che parliamo del settore del pomodoro, in cui il provvedimento imposta un percorso con tutti i passaggi, dalla produzione alla trasformazione fino al prodotto finito, sia che parliamo del settore del riso, di cui si sostengono gli sviluppi di miglioramento genetico, del rapporto tra prodotto e territorio e paesaggio, del miglioramento dell'informazione per i consumatori. Si affrontano settori consolidati e tradizionali dell'agroalimentare italiano, ma anche settori che stanno emergendo, pur in piccole quantità, ma che arricchiscono il patrimonio italiano. Mi riferisco all'articolo che concerne le birre artigianali, la definizione di birra artigianale che andrà ancora approfondita ed una regolamentazione dei piccoli birrifici che tenga insieme tracciabilità e semplificazione, cioè regole compatibili con le piccole dimensioni. Ecco, credo che l'importanza di questo provvedimento stia nei temi che affronta, ma anche in un nuovo approccio, che tiene sullo stesso piano le grandi dimensioni, le riforme strutturali generali, ma anche la definizione e la regolamentazione delle produzioni emergenti, di piccola nicchia. Riforme generali e regolamentazioni delle specificità: è l'approccio che credo debba avere il nostro Paese parlando non dell'agricoltura, ma delle agricolture, diverse, riconosciute e certificate. Credo che si possa affrontare una nuova fase, che vi sia una nuova opportunità per le nuove generazioni e quindi esprimo tutta la soddisfazione di essere arrivata alla fine di questo percorso, perché conferma che questo Governo, come come mai era successo prima, ha messo al centro l'agricoltura e la sua modernizzazione in questo nuovo tempo, e questo è un cambiamento di grandissimo significato.

intervento avrei proprio preferito non farlo, perché con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo, a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Ieri abbiamo saputo che l'elenco delle donne vittime di femminicidio si è allungato di una unità. Micaela Masella è morta il 12 giugno per mano del marito da cui era separata da due anni, che ha provocato l'esplosione dell'appartamento in cui vivevano lui, Micaela e due figlie. Nell'esplosione sono morti Micaela Masella e una coppia di vicini. Le due figlie sono ferite e ancora ricoverate al Niguarda. Il marito ha confessato ieri che ha staccato il tubo del gas in casa perché non sopportava l'abbandono della moglie che, dopo due anni di separazione, in cui non aveva ancora interrotto la convivenza, aveva deciso di andare a vivere con un nuovo compagno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'onore tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo, un *raptus*. Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità, in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che determinano l'asimmetria. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Che cosa non ha funzionato nel piano per la protezione di Micaela Masella? Quali misure preventive andavano messe in campo per evitare una tragedia del genere? Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza.

si avvicina un disastro ben maggiore. Secondo le ultime analisi di Bloomberg, le banche cinesi richiederanno entro due anni al massimo, fino a 3.000 miliardi di dollari di ricapitalizzazione. Una bomba cinque volte più devastante del caso Lehman Brothers. Il Governo cinese dovrà svalutare lo yuan almeno del 30 per cento e spingere, spingere le esportazioni. E si stanno attrezzando: alla via della seta ferroviaria transasiatica, si aggiunge quella marittima, attraverso il canale di Suez recentemente raddoppiato, che si completa col progetto del porto *off-shore* di Venezia. Un'opera che agli italiani non serve, ma al presidente dell'Autorità portuale Costa sì, e ai cinesi pure. Tra Prato, Padova e Milano è consolidato un distretto industriale, ma anche una rete distributiva per l'invasione delle merci cinesi. I tumulti di Sesto Fiorentino sono in linea con la creazione di uno Stato nello Stato, in violazione sistematica delle regole del Paese ospitante: dall'elusione fiscale alla giustizia sommaria. Un controllo di *routine* è stato ostacolato con violenza, con il coinvolgimento di una associazione, il Cervo bianco, dedita a pestaggi e intimidazioni, che ha ai vertici condannati per omicidio e fatti di prostituzione. Come è possibile, ministro Alfano? Risponda alla mia interrogazione. Questi "*vigilantes*" proteggevano interessi di imprenditori cinesi, che hanno troppo denaro contante: lo dice il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Ogni anno attraverso i *money transfer* passano in Cina 1,7 miliardi; in Veneto, secondo uno studio della Camera di commercio, sono molto più dei redditi dichiarati. proteggono una fitta rete di ditte individuali, che cambiano ragione sociale prima di dover depositare i bilanci, che producono o importano prodotti tossici per la salute e continuamente oggetto di sequestri. È cieco o in malafede chi non vede la strategia di uno Stato che fintamente ha abbracciato il mercato, ma agisce secondo logiche stataliste di derivazione comunista, uno Stato che, invece di abbracciare i diritti umani e la protezione dell'ambiente, ne fa scempio, per avere un indebito vantaggio sull'Europa. Che la Cina si possa considerare una economia di mercato è ridicolo. Ci pensi il Partito Democratico, troppo morbido in Europarlamento: a quali interessi sta aprendo la porta? Ci pensi il ministro Alfano, che ha fatto pattugliare Roma e Milano a poliziotti cinesi nelle loro uniformi, come se a valere non fosse la nostra legge e fossimo disposti ad una cessione di sovranità nazionale. Le nostre Forze dell'ordine sono bloccate da tagli e tagli, mentre il loro sistema può pagare lautamente studi legali e commercialisti compiacenti. Non c'è nulla di segreto in questo: questa guerra di conquista commerciale è oggetto di articoli e pubblicazioni internazionali. Signori, o apriamo gli occhi o chiuderanno le nostre fabbriche, per sempre.